Città di Castello e tutta l'Umbria sono in lutto, così come ieri lo sono stati il Veneto e la città di Vicenza, per la tragica morte

di persone che perdono il controllo di se stesse. Questo giovane ufficiale superiore, proveniente dall'alta Valle del Tevere, da un'antica famiglia, già ricca di sacrifici, con un grande *curriculum* di servigi resi alla società, nel tentativo generoso di salvare delle vite e di scongiurare atti di pazzia si è visto esplodere dei colpi di arma da fuoco che lo hanno freddato.

La ringrazio, signor Presidente. a nome mio personale e dell'intera Assemblea che ho l'onore di presiedere, mi associo al dolore dei familiari e dell'Arma per questo grande tributo reso a tutela dell'ordine pubblico e della legalità.

Il motivo per il quale è stato modificato il calendario è evidente. La maggioranza ritiene che tra qualche mese le vicende del Presidente del Consiglio si presenteranno al Paese più sfumate e meno pericolose. L'idea è che il trascorrere del tempo possa addormentare l'opinione pubblica. In nessuna democrazia evoluta, tranne che nell'Italia del 2009, avrebbe senso presentare documenti parlamentari dal contenuto analogo a quello delle due mozioni. Da noi è necessario. A tre mesi dall'inizio di uno scandalo che ha avuto un'eco mondiale, il Parlamento non se ne è mai occupato. Mai il Governo ha risposto alle interrogazioni, né ha trovato altro modo per informare Camera e Senato. Le mozioni Soliani e Zanda sono anche conseguenza di questa censura del Governo. Il loro senso politico è chiaro. La prima impegna il Governo al rispetto della stampa internazionale. La seconda a dire la verità e a non mettere in pericolo la sicurezza nazionale con comportamenti imprudenti. Non mi sembrano richieste stravaganti o eversive. Riguardano fatti gravi, avvenimenti sconcertanti, che hanno offuscato la credibilità dell'Italia nelle settimane e nei mesi che hanno preceduto e preparato il G8. La mozione Soliani è diretta ad impedire il ripetersi di quel che è già realmente accaduto prima del G8. Il Governo Berlusconi rispetta la stampa solo quando descrive i fatti in modo gradito o li commenta con favore. La strapazza o la insulta quando dissente, quando avanza obiezioni, quando si oppone. Il Governo vorrebbe molto semplicemente che le notizie sgradite non venissero pubblicate. Quando accade, si risente. Il Partito Democratico ritiene che il pieno rispetto della stampa, stampa, specie di quella più critica, sia un principio fondativo di tutte le democrazie moderne e chiede al Senato di confermare questo indirizzo. La mozione a mia prima firma, invece, pone la questione del rilievo pubblico dei comportamenti di chi governa il Paese, anch'essa emersa prima del G8. La mozione è stata variamente interpretata, non sempre rispettandone il significato, talvolta stravolgendone il senso. Debbo, quindi, essere chiaro e indicare non solo quel che la mozione propone, ma anche quel che non ha inteso sostenere. A nessuno dei firmatari è mai passata per l'anticamera del cervello l'idea di porre il tema della moralità privata degli uomini politici, della loro fedeltà coniugale, delle loro abitudini sessuali, dei loro appetiti di ogni genere e specie. Se non viene violata la legge, queste questioni non possono e non debbono interessare il Parlamento. Anche il tema del decoro dei comportamenti di chi ci governa, pur così rilevante per l'opinione pubblica mondiale, non è l'obiettivo fondamentale della mozione. Se oggi siamo costretti a prospettare la necessità di regole minime di decoro è perché è stato travolto ogni limite di decenza, non c'è più nessuna misura, sono emersi così tanti e così smodati eccessi che i comportamenti privati hanno finito col condizionare lo stesso funzionamento delle istituzioni. Il problema di porre un limite all'indecorosità dei comportamenti non lo pone l'opposizione, ma l'evidenza delle cose. Ieri ed oggi sono stati resi noti colloqui del Presidente del Consiglio che confermano ancora una volta questa evidenza al di là di ogni ragionevole dubbio. Peraltro, anche nei rapporti parlamentari sono stati superati tutti i limiti di una corretta supremazia della maggioranza nei confronti dell'opposizione. La decisione di tenere fuori dal dibattito parlamentare sino a settembre fatti straordinariamente rilevanti per la sicurezza nazionale costituisce una prevaricazione dei diritti dell'opposizione e conferma quanto oggi la destra italiana si consideri onnipotente allorché si tratta di tutelare i propri interessi politici. L'imposizione ripetuta della forza parlamentare per condizionare il procedimento legislativo con decreti-legge, voti di fiducia, maxiemendamenti, leggi *omnibus* ed oggi persino con una forzatura al calendario è segno solo di mera potenza numerica, non di intelligenza politica, non di sensibilità per gli interessi generali del Paese, non di lungimiranza parlamentare. Vi sono, infatti, due aspetti di quanto è emerso dalla condotta del Presidente del Consiglio sui quali, se la maggioranza fosse capace di maggiore responsabilità, il Senato dovrebbe pronunciarsi immediatamente. La prima questione è se il Presidente debba impegnarsi a dire sempre e comunque la verità. Gli ultimi scampoli di conversazione resi noti ieri ed oggi sono lì a dimostrare quanto ci sia bisogno che chi governa il nostro Paese dica la verità. Anche nel dire il vero o il falso il presidente Berlusconi ha superato ogni limite consentito. Non esiste al mondo alcuna Nazione dove la menzogna dei governanti non corrompa pericolosamente la società e le istituzioni. In una democrazia evoluta la legittimazione politica a governare deve essere confermata giorno per giorno. Il presidente Berlusconi lo sa bene e diffonde quotidianamente sondaggi fatti in casa. Sinora, però, i suoi uffici non hanno mai promosso sondaggi seri per sapere se gli italiani vogliono un Capo del Governo che dice sempre e comunque la verità o se si accontentano che la dica solo quando gli conviene. Ed è su questo punto che la mozione chiede che si esprima il Senato. La seconda questione è ancora più rilevante. Riguarda i comportamenti del Primo Ministro, compresi quelli della sua vita privata. La mozione chiede che i comportamenti di chi ci governa vengano improntati alla prudenza necessaria per non mettere in pericolo, nemmeno potenzialmente, la sicurezza nazionale. Abbiamo saputo di feste con numerose e incontrollate ospiti. Abbiamo saputo e visto gli effetti di registratori e macchine fotografiche. Abbiamo appreso da un amico del Presidente che ad un certo punto, durante le feste, arrivava il maggiordomo con una pila di *dossier* che il Presidente doveva firmare o esaminare. Non conosciamo quale fosse il contenuto dei *dossier*, ma conosciamo l'ampiezza delle competenze del Primo Ministro e la necessità che abbia continuo accesso a informazioni anche segretissime sul piano nazionale e internazionale. Il Senato dovrebbe mostrare grande preoccupazione nell'apprendere che carteggi governativi giravano negli stessi ambienti dove avevano libero accesso personaggi incontrollati. Anche qui gli stessi comportamenti: il Presidente sembra non rendersi conto che per un uomo di Stato l'imprudenza ha limiti ben precisi. Davanti a queste informazioni il minimo che può succedere è che le cancellerie dei Paesi della NATO, dei nostri alleati e di quelle potenze con cui abbiamo buoni rapporti stiano valutando quali informazioni sensibili possano essere ancora portate senza rischi a conoscenza del Governo italiano. In altre democrazie quel governante che mettesse a rischio in questo modo gli interessi del suo Paese perderebbe immediatamente la fiducia del Parlamento. A garanzia della sicurezza nazionale chiedo che il Senato venga rassicurato sul fatto che questi comportamenti sono cessati e informato su quali rischi l'Italia ha corso o sta ancora correndo. Ecco perché chiedo che le due mozioni vengano discusse subito. Il senatore Gasparri ha accusato ripetutamente l'opposizione di scorrettezza. Ad altri senatori risponderei per le rime, a Gasparri no. Ci ha abituato a questi modi. Ma le sue minacce non ci impressionano. Credo che non gioverebbe al presidente Berlusconi un dibattito parlamentare che, come lo stesso senatore Gasparri ha più volte minacciato negli ultimi giorni, veda affrontati i problemi della sicurezza nazionale derivanti dai comportamenti presidenziali in parallelo con il caso di quel Bianchini che la nostra polizia accusa di delitti sessuali schifosi. È un accostamento che non vorrei veder fatto in Senato. Il Presidente della Camera, onorevole Fini, ha ammonito come oggi sia «a rischio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni». Il presidente Fini ha ragione. Ma i cittadini non hanno torto a sfiduciare le istituzioni quando la maggioranza arriva a minacciare pubblicamente ritorsioni parlamentari per evitare di discutere della sicurezza nazionale e della dignità del nostro Paese. *(Applausi

la modifica del calendario che era stato concordato e non lo abbiamo fatto per ragioni di metodo. In primo luogo, perché credo che quando il tema è sostanziale, cioè c'è una diversità di vedute sul piano politico in merito ad alcune questioni, non ci si può trincerare dietro un giudizio di attinenza o non attinenza all'oggetto della mozione di natura parlamentare. Nel caso in esame le mozioni presentate dai colleghi dell'opposizione - come ho detto subito in occasione della Conferenza dei Capigruppo - quest'ultima mozione - da noi non condivisa e, se iscritta all'ordine del giorno e discussa, destinata certamente un'attinenza ce l'hanno. Ma delle mozioni presentate da Gruppi dell'opposizione non possono essere cancellate dal calendario un'ora prima della discussione in

l'idea di non accedere ad una discussione parlamentare su un tema purtroppo di attualità (tema che, per la verità, se il Presidente del Consiglio, come aveva annunciato, avesse

con l'aggiunta che si cerca di far passare tale iniziativa come censoria perché la maggioranza rifiuta ad un Gruppo parlamentare di opposizione di discutere una mozione, indipendentemente dal contenuto della stessa, su cui

un codice che vale solo per alcuni che sono investiti di una funzione pubblica e non per altri. Questa è una mozione che ha ad oggetto alcune questioni specifiche e deve avere il coraggio di affrontarle in maniera specifica. Nel caso di specie, dal nostro punto di vista, una mozione una mozione di questa natura, o qualsiasi altra iniziativa avente ad oggetto un'inchiesta parlamentare, anziché cercare di scrivere un codice di deontologia parziale, avrebbe introdurre alcuni elementi che nel dibattito su questa vicenda non sono stati introdotti. Penso, ad esempio, alla circostanza che Villa Certosa è coperta da segreto di Stato per un'espressa richiesta del Governo del tempo, nella legislatura 2001-2006, e che quindi dovrebbe essere soggetta a regole di accesso e di pubblicità che non sono quelle che oggi leggiamo sui giornali. Stesso discorso riguarda le altre residenze del Presidente del Consiglio, l'accesso alle quali deve essere per natura assolutamente limitato. Un'inchiesta parlamentare che avesse ad oggetto queste vicende specifiche, che riguardasse in maniera specifica interessi della sicurezza dello Stato potrebbe dal nostro punto di vista trovare ingresso nel dibattito parlamentare. Una mozione molto generica, che rischia di essere un'arma a doppio taglio, non è per noi condivisibile. non preclude però che la circostanza debba essere oggetto di un dibattito e che oggi si sia leso un diritto della minoranza: quello di poter introdurre nel confronto parlamentare

perché riteniamo che rientri nelle peculiarità del Parlamento affrontare temi di enorme interesse il fine di impegnare il Governo su problematiche non estranee alla salute della Repubblica.

il che significa che il Parlamento è il luogo centrale della democrazia, del dibattito e delle discussioni. E quando in un'Aula del Parlamento si vuole introdurre il discorso sul rispetto che che si deve garantire nell'applicazione concreta dell'articolo 21 della Costituzione (dedicato all'esercizio del diritto di cronaca e di critica) si affronta un tema fondamentale della nostra democrazia. Non è un tema estraneo. Quando nella mozione con cui si voleva impegnare il Governo vengono affrontati i temi del decoro, della sicurezza, della sobrietà e della riservatezza,

Pensiamo veramente che non debba impegnarsi il Governo, né debba essere motivo di discussione quanto è avvenuto e continua ad avvenire in queste ore? Un Presidente del Consiglio che ad una persona estranea, parlando del G8 (parlando del G8, non di altre cose), «Nei prossimi giorni presiederò il G8, poi diventerà il G14 ed io guiderò la politica economica dell'80 per cento del mondo perché sono insuperabile» non è un tema da discutere? Non riguarda il Parlamento sentire il Presidente del Consiglio che scandisce: «Insuperabile, nessuno mi può battere, dirigerò l'economia del mondo»?

Caro senatore Zanda, poiché lei prima diceva che invece noi non le vogliamo discutere per allungare i tempi affinché l'opinione pubblica in qualche modo resti addormentata sul tema, le dico che all'opinione pubblica della sua mozione non gliene frega niente: gliene importa zero della vita privata del *Premier*.

su questi temi è inutile sprecare troppe parole, che gli sciacalli siano più simpatici di chi, in questo momento, cerca solo di strumentalizzare gli atti del nostro Governo a danno dell'intero Paese. Presidente, anch'io, senza mettere in discussione la democrazia parlamentare e senza scomodarla, in quanto non credo ne valga la pena, vorrei tornare su un punto che è molto semplice. Alla Conferenza dei Capigruppo era stata decisa la calendarizzazione di mozioni sul G8 e sulle sue conclusioni.

ma c'era una ragione di buon senso che per un *gentlemen's agreement* tra maggioranza ed opposizione è stata fatta valere, per cui quella decisione è stata assunta prima che le conclusioni del vertice de L'Aquila fossero note, e questo anche a riprova della buona volontà da parte della maggioranza, dal momento che nessuno sapeva quello che le mozioni dell'opposizione riconoscono e cioè che quel G8 sarebbe stato un successo. Si è ritenuto, tuttavia, che fosse un dritto dell'opposizione chiedere quella discussione e un diritto di quest'Assemblea

ha presentato una mozione sulle conclusioni del G8, di cui ora sentiremo l'illustrazione, ma quando si è trovata di fronte ad altri documenti che trattano (come abbiamo sentito dall'esposizione del collega Zanda,

e cioè il problema della stampa internazionale, il problema del rapporto tra moralità privata ed etica pubblica ed il problema della sicurezza dello Stato, la maggioranza, si è trovata a non aver presentato alcun documento su queste materie. prerogativa dell'opposizione che è quella di poter far discutere i documenti che vuole, ma fino a prova contraria in democrazia c'è anche la prerogativa della maggioranza di poter intervenire

il presidente Gasparri non ha fatto altro che riprendere alcune considerazioni avanzate da un senatore del suo Gruppo all'interno di un dibattito in vista del congresso del suo partito. Questo è l'atto di irresponsabilità che lei ora gli rimprovera. Si rivolga a colui il quale queste argomentazioni ha proposto.

per poter intervenire in maniera documentata. A questo proposito nessuno sta pensando di attentare alla centralità del Parlamento, né tanto meno di mettergli il bavaglio. Io non parlerò non parlerò di inganno, ma i margini su cui si gioca il confronto tra maggioranza e opposizione, in questo caso, sono stati utilizzati un po' troppo liberamente.

niente di più, niente di meno. Nessuno, da questa parte, accetta lezioni sulla responsabilità, perché è troppo facile dichiararsi responsabili sulle agenzie

*(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo richiesto e fortemente voluto questo momento di discussione nell'Aula del Senato perché potesse essere un'occasione di riflessione meditata, ma anche e soprattutto un momento di impegno sui temi della sicurezza ferroviaria. Una sicurezza che il tragico evento di Viareggio ha riproposto con violenza agli occhi dell'opinione pubblica in tutta la sua drammatica

signor Presidente. Come dicevo, abbiamo richiesto e fortemente voluto questo momento di discussione nell'Aula del Senato affinché potesse essere un'occasione di riflessione meditata, ma anche e soprattutto un momento di impegno sui temi della sicurezza ferroviaria. Una sicurezza che il tragico evento di Viareggio ha riproposto con violenza agli occhi dell'opinione pubblica in tutta la sua drammatica evidenza. Abbiamo denunciato - in vero non da soli - più di una volta, ancora prima dei fatti di Viareggio, che sul tema della sicurezza, nei sistemi di trasporto... No, la sicurezza non è un tema di grande interesse, anche se a Viareggio ha prodotto qualche risultato negativo. FILIPPI Marco *(PD)*. Provo a ripetere. Abbiamo denunciato - invero non da soli - più di una volta, ancora prima dei fatti di Viareggio, che sul tema della sicurezza, nei sistemi di trasporto ferroviario, occorreva alzare il livello di attenzione perché il livello di guardia si era pericolosamente abbassato. Lo abbiamo sempre fatto con compostezza, senza strumentalizzare fatti o circostanze, che abbiamo però denunciato con la massima determinazione, cosa che abbiamo intenzione di continuare a fare, consapevoli del fatto che il nostro compito e la nostra ambiziosa missione non si esauriscono certo con una discussione alta nelle massime sedi istituzionali. *(Brusìo).*

che abbiamo però denunciato con la massima determinazione, cosa che abbiamo intenzione di continuare a fare, consapevoli del fatto che il nostro compito e la nostra ambiziosa missione non si esauriscono certo con una discussione alta nelle massime sedi istituzionali e con l'assunzione di solenni impegni che poi spesso, come da tradizione, rimangono lettera morta. No, rivendichiamo per noi e per il Parlamento un'altra funzione: quella che, finito il momento del lutto e del dolore più acuto (non dimenticando che c'è ancora chi lotta per scampare alla morte), individua il momento del fare per riparare ciò che c'è da riparare, ma soprattutto per far sì che eventi simili non si debbano più ripetere. Perciò, occorre avere la massima attenzione a tutta la filiera della sicurezza, una catena la cui affidabilità e garanzia si calcolano come per tutte le catene sull'anello più debole e non certo sulla maglia più solida e forte. I fatti di Viareggio - a mio parere - ci dicono che siamo in presenza di almeno tre anelli più deboli degli altri, per i quali occorre non indugiare ma procedere celermente con gli atti e i provvedimenti necessari. Il primo anello debole è costituito dalla lunghezza della catena di controllo della sicurezza: tanto più lunga è la catena dei soggetti preposti al controllo e tanto è più probabile che un controllo non venga effettuato a dovere o addirittura non venga fatto per niente.

I fatti di Viareggio - a mio parere - ci dicono che siamo in presenza di almeno tre anelli più deboli degli altri, per i quali occorre non indugiare ma procedere celermente con gli atti e i provvedimenti necessari. Il primo anello debole è costituito dalla lunghezza della catena di controllo della sicurezza: tanto più lunga è la catena dei soggetti preposti al controllo e tanto più è probabile che un controllo non venga fatto a dovere, o che addirittura non venga fatto per niente. Questo è l'anello, tra tutti, che si è rivelato decisamente più debole. E legato a questo anello vi è il sistema delle certificazioni dei vari soggetti, che è apparso sostanzialmente un artificio amministrativo privo di efficacia operativa e privo delle necessarie sanzioni, che costituiscono il principale deterrente ai comportamenti omissivi ed elusivi. Nel caso di specie, ovviamente la magistratura ordinaria è chiamata a fare il suo corso; noi speriamo presto e bene. Voglio però evidenziare una particolarità che abbiamo segnalato nella nostra mozione e che rappresenta un paradosso davvero incredibile. Il livello dell'attenzione sulla sicurezza che la normativa prevede nei luoghi di attività e di stoccaggio delle merci pericolose inspiegabilmente si abbassa durante il loro trasporto e nei luoghi di trasbordo e di stoccaggio temporaneo, proprio dove più alto è il rischio di incidenti. Occorre in questo senso che i principi contenuti nella direttiva "Seveso 2" per le aree a rischio di incidente rilevante, probabilmente analoghi a quelli della più recente direttiva comunitaria, rappresentati nella loro essenza dall'analisi e della certificazione dei rischi e dalle procedure di informazione per la messa a conoscenza delle pubbliche autorità, siano immediatamente estesi anche a questi ambiti di attività. Il secondo anello debole è costituito dal quadro normativo esistente, particolarmente carente nel recepimento delle direttive comunitarie emanate, aspetto, questo, che si fa particolarmente delicato nell'attuale processo di liberalizzazione dei sistemi di trasporto ferroviario, merci e passeggeri, soprattutto quando le stesse direttive vengono recepite dagli Stati membri con differente tempistica e con libera interpretazione. Gli aspetti di reciprocità rischiano in questo senso di compromettere, al contempo, sia i livelli di sicurezza che di concorrenza che le liberalizzazioni sono, invece, chiamate a perseguire. Su questo punto le mozioni sono sostanzialmente sovrapponibili, indicando con precisione le cose non fatte e da fare, ma anche quelle che possono essere ulteriormente fatte, perché la sicurezza non è una condizione che si raggiunge una volta per tutte, e dove il meglio non è nemico del bene. Il terzo anello debole è la costituzione di un soggetto autonomo e indipendente deputato ad assicurare gli standard di sicurezza, così come previsto dalla direttiva 2004/49/CE, recepita con il decreto legislativo n. Su questo aspetto che la nostra mozione pone al centro, ma che è presente, comunque, anche in tutte le altre, occorre al più presto rendere operativa l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria evitando ulteriori, inutili e dannose lungaggini burocratiche, resistenze corporative o sabotaggi striscianti. Insomma, per realizzare un sistema di trasporto ferroviario che deve essere regolato, liberalizzato, efficiente e sicuro, occorre prioritariamente realizzare un sistema fatto di competenze e titolarità chiare e ben definite. Un sistema fatto, cioè, di soggetti che in autonomia e responsabilità, in regime di libera concorrenza, intendono offrire servizi, ma anche di soggetti chiamati a fare da arbitri con l'indipendenza e l'autorevolezza che derivano loro dall'esercizio degli effettivi poteri previsti, nell'esclusivo interesse dei cittadini e a garanzia di una sicurezza che non può essere oggetto di nessuna negoziazione. A questo riguardo è confortante la presentazione di mozioni i cui testi, per quanto si differenzino nel linguaggio e nel taglio conferito, sono in larga parte condivisibili e nelle loro parti dispositive ampiamente omogenee. Verrebbe da dire che abbiamo tutti chiaro ciò che c'è da fare e al Governo viene pertanto chiesto di provvedere con la massima celerità. di aggiungere a corollario anche alcune sottolineature volutamente non presenti nel nostro testo, ma che ho visto contenute in altri e che voglio anch'io enfatizzare nel dibattito.

il frutto di un'effettiva ottimizzazione delle risorse. Noi, comunque, vigileremo e terremo alta l'attenzione, come è nostro dovere fare. Desidero sottolineare anche la questione del clima aziendale, che nelle ferrovie, proprio sulla sicurezza, ha mostrato, talvolta, il volto incomprensibilmente più duro e foriero di un messaggio implicito che sulla sicurezza condanniamo nella maniera più ferma. Non si alza il livello di sicurezza, né quello effettivo né quello percepito, con le punizioni o con i provvedimenti disciplinari esemplari, come è avvenuto proprio per i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza. Alle denunce dei lavoratori, anche quando queste fossero inesatte, si risponde con maggiore trasparenza e maggiore informazione, proprio su quelle scelte che l'azienda ha fatto, probabilmente nel giusto, ma che possono presentare profili contraddittori nell'opinione prevalente dei lavoratori e che proprio per questo hanno bisogno di maggiore e non di minore informazione, di massima umiltà nella fermezza delle decisioni da assumere, e non con gesti sprezzanti per un coraggio che sulla materia della sicurezza davvero non è richiesto. *(Applausi

quando accadono incidenti ferroviari come quello avvenuto a Viareggio, ci sentiamo tutti impegnati a dare risposte a domande del tipo: si poteva evitare? Cosa si può fare per evitare che accada di nuovo?

vorrei che almeno ora si continuasse a non fare riunioni nell'emiciclo. consentirebbero di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza nel trasporto ferroviario del nostro Paese e degli altri Paesi dell'Unione europea. Registro anch'io, con indubbia soddisfazione

sull'impegno che vogliamo chiedere con forza al Governo affinché si faccia davvero un salto di qualità anche in questo settore. La nostra analisi parte dalla constatazione che nel settore dei trasporti ferroviari l'incidentalità mortale è tra le più basse d'Europa, che i livelli di sicurezza delle ferrovie italiane sono allineati con quelli delle principali reti comunitarie, che i sistemi tecnologici nel campo della sicurezza sviluppati in Italia sono tra i più moderni d'Europa, anche a seguito di importanti investimenti realizzati proprio negli ultimi dieci anni, e che il treno rappresenta ancora oggi il mezzo più sicuro e sostenibile per il trasporto sia di persone, che di merci, pericolose e non. Tuttavia, l'esame di quanto accaduto a Viareggio e soprattutto delle procedure praticate in osservanza delle direttive europee e delle norme esistenti nel nostro Paese e negli altri Paesi dell'Unione europea la valutazione attenta di come concretamente si muovono gli operatori del settore in osservanza di dette procedure ci hanno convinto dell'esistenza di lacune e contraddizioni che vanno al più presto superate e rimosse, se vogliamo davvero elevare le condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario anche in Italia. Infatti, ad oggi: non esiste, neanche a livello comunitario, una direttiva precisa in materia di certificazione delle officine preposte alla manutenzione ed alla revisione del materiale rotabile; il sistema delle revisioni a tempo del materiale rotabile destinato al trasporto merci è obsoleto o quantomeno insufficiente, considerato che la liberalizzazione e l'utilizzo dei carri merci si è sviluppato in modo davvero intensivo in questi ultimi cinque anni; il sistema delle revisioni risulta essere disomogeneo tra i vari Paesi d'Europa anche per quanto riguarda le competenze e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nel processo di manutenzione. Per questi motivi, signor Presidente, riteniamo si debba intervenire, si debba intervenire, a livello sia europeo che di normativa nazionale, per evitare che la costante apertura del mercato ferroviario all'interno di un processo di liberalizzazione che non può arrestarsi, ma che deve essere sempre più controllato e regolato, comporti ritardi e applicazioni eterogenee tra Paese e Paese nel settore della sicurezza del trasporto ferroviario. Per questo, ci facciamo portatori di una richiesta che impegni l'Unione europea all'emanazione di una norma volta a stabilire criteri di certificazione comune a tutti gli Stati membri per l'individuazione di officine di manutenzione certificate dalla Unione

verifica del chilometraggio e del peso, al posto della verifica temporale, quale fattore discriminante nel processo di revisione dei veicoli. si debbano compiere a livello nazionale alcune azioni da parte del Governo, ben indicate nella nostra mozione, relative alla piena attuazione delle normative internazionali e comunitarie, anticipando i termini di recepimento della ratifica della convenzione del COTIF, dell'attuazione della direttiva 2007/57/CE dell'Unione europea e dell'attuazione con decreto legislativo della normativa europea relativa al trasporto di merci pericolose su ferro. vorremmo il completamento da parte dei Ministeri competenti del contesto regolamentare, organizzativo e gestionale, che consenta all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di meglio assicurare l'esercizio delle missioni e delle responsabilità ad essa legislativamente attribuite.

Suggeriamo questa iniziativa perché dai quotidiani risulterebbe che le Ferrovie dello Stato rifiuterebbero di indennizzare le famiglie dei caduti e le persone che hanno avuto danni sensibili in tale occasione. I soggetti titolari dei carri ferroviari fanno altrettanto, in assenza di una

onorevoli senatori, troppo spesso nella nostra Italia sono necessarie sciagure come quella che si è consumata a Viareggio nella notte del 29 giugno per indurci a riflettere e ad assumere provvedimenti rispetto a problematiche che richiederebbero, al contrario, una costante attenzione per evitare drammi analoghi alla recente catastrofe ferroviaria che ha dilaniato intere famiglie e ferito nel cuore una città. Il tema della sicurezza in genere dovrebbe essere costantemente all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, per creare quella cultura diffusa in materia che è presupposto imprescindibile per evitare incidenti di ogni genere e grado nei più disparati settori. Al contrario, si riflette sul tema della sicurezza sempre *a posteriori*, quando si debbono contare i morti a fare la stima dei danni. Questo atteggiamento non è più accettabile. A livello europeo l'Italia è tra quei Paesi ove si verificano meno incidenti ferroviari gravi: 130, dopo l'Inghilterra che si attesta a 110 e prima della Germania, che ne conta 319, e della Francia con 413. Effettivamente, come si evince dal rapporto annuale sulla sicurezza della circolazione dei treni per il 2007, redatto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, risulta in diminuzione il totale degli incidenti ferroviari, che passa dai 134 incidenti del 2005 ai 121 del 2007. Tuttavia, questo *trend* positivo sembra essersi interrotto, se consideriamo che quest'anno, in soli venti giorni, se ne sono verificati ben precisamente il 19 maggio a Sesto Calende, il 22 giugno a Vaiano, il 21 giugno a Pisa e il 29 a Viareggio con la tragedia di cui tutti siamo stati testimoni. Non è un caso che ben tre dei quattro incidenti hanno interessato treni merci. Risale, peraltro, a pochi giorni fa, martedì scorso, 14 luglio, l'ennesimo episodio. I vigili del fuoco sono stati impegnati a mettere in sicurezza un'area della stazione centrale di Messina, giacché un convoglio che trasportava azoto liquido perdeva gran parte del suo carico a causa del cedimento della valvola di sicurezza imputabile ad un cambio di pressione dovuto alle alte temperature del periodo. Nella stazione di Messina la situazione è particolarmente grave per il permanere di convogli merci per lungo tempo nella stazione, visto il ridotto numero di navi RFI impegnate sullo Stretto. A questo punto, appaiono necessarie delle riflessioni, con particolare riferimento agli effetti che il processo di liberalizzazione ha prodotto sia a livello nazionale che a livello europeo. In Italia, in ossequio alla disciplina comunitaria, si è andato avviando tale processo che, non pienamente compiuto, ha determinato una situazione di sostanziale monopolio della mobilità ferroviaria in capo a Trenitalia spa. Da sola essa effettua il 97,59 per cento del volume del traffico totale sulla infrastruttura ferroviaria. Questa condizione ha fatto e fa prevalere nell'azienda una logica di *business* che induce a tagliare tutti i servizi non redditizi, privilegiando in tale ottica l'Alta velocità a danno del cosiddetto servizio universale. Questa politica orientata al profitto ha portato in pochi anni a ridurre la dotazione organica delle Ferrovie da 220.000 a 83.000 unità, a tagliare circa 8-9 milioni di chilometri-treno da Ancona in giù e da Napoli in giù. Le ricadute di questa scelta si rifletteranno su Regioni come la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania. Si è proceduto, inoltre, a ridurre del 50 per cento i treni a lunga percorrenza e si è abbandonato quasi completamente il settore merci, che versa in condizioni di A tal proposito, si è chiuso sostanzialmente il trasporto ferroviario merci per la Sardegna, negando la cosiddetta continuità territoriale e si procede a contrarre quello sullo Stretto di Messina. L'entrata a regime dell'Alta velocità ha inoltre sviluppato criticità sui nodi ferroviari, aggravando la già drammatica situazione della regolarità e puntualità del trasporto pubblico locale, carente di *comfort* e igiene, come denunciano i comitati dei pendolari. Si sta delineando, insomma, un'Italia a due velocità, una che può correre in competizione con l'aereo e l'altra che resterà sempre più arretrata, ampliando le differenze sociali ed economiche del Paese. Noi non possiamo avallare questa politica. A nostro avviso, in ossequio al principio costituzionale che sancisce la libertà di circolazione per tutti, le ferrovie devono essere uno strumento attraverso cui garantire coesione sociale e sviluppo economico per tutto il Paese La prevalente logica di *business* ha, inoltre, portato a penalizzare fortemente settori come la manutenzione e, quindi, la sicurezza. Il cosiddetto materiale rotabile ha una media di 20 anni di servizio, 10 in meno quello dell'Alta velocità; l'età media del parco carri in esercizio è di 24 anni tra il 2008 e il 2009; ne sono stati demoliti più di 5.000 in quanto non idonei. Nel corso di quest'anno 7.000 degli attuali 16.000 chilometri di infrastruttura ferroviaria nazionale potrebbero essere sottoposti ad un regime manutentivo e di esercizio più economico dell'attuale, aggravando il già elevato rischio, in tale settore, di infortuni sul lavoro. A causa del prevalere di una politica di esternalizzazione, l'attività manutentiva è affidata in piccola parte al gruppo Ferrovie dello Stato (soprattutto sui rotabili) e per la gran parte ad imprese private. Le lavorazioni esterne non sempre risultano giustificate sotto un profilo economico e di affidabilità. Infatti, le officine private esterne difettano di certificazioni e qualificazioni di verificatori indipendenti di sicurezza. Gli allarmi inutilmente lanciati in questo campo hanno fatto divenire quella di Viareggio l'ennesima tragedia annunciata. A questa situazione si aggiungano i tagli che questo Governo ha effettuato: nel capitolo dedicato alla sicurezza si passa da 15 milioni del rendiconto 2007 a nessuna previsione nell'assestamento 2009; nel capitolo 7122, relativo agli investimenti per sviluppare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie, si passa da 3.511 milioni del rendiconto 2007 a 2.362 2.362 milioni dell'assestamento 2009. Quando si parla di infrastrutture le classifiche internazionali sono impietose: l'ultima graduatoria stilata dal *World Economic Forum* ci piazza al 54° posto su 134 Paesi. Ancora peggio se si analizza la qualità delle opere, perché scivoliamo addirittura al 73° posto. Non è prevista alcuna provvidenza a favore del settore sicurezza neppure nella cosiddetta manovra estiva all'esame del Parlamento. Un'ulteriore riflessione va fatta in merito al processo di liberalizzazione della mobilità ferroviaria in Europa, cui non è seguito un processo di integrazione europeo dei controlli. Mentre fino a poco tempo fa infatti vi era un unico soggetto, cioè le Ferrovie dello Stato, che gestiva servizio e sicurezza, oggi il processo di liberalizzazione ha comportato come primo effetto la separazione tra gestore della rete e gestori dei servizi. Attualmente, a fronte di un unico gestore della rete, abbiamo circa 30 imprese ferroviarie, tra cui Trenitalia in posizione di monopolio, e i proprietari dei carri. A breve avremo più gestori della rete perché vi saranno i gestori delle reti regionali. A costoro vanno aggiunti i costruttori, le officine e gli organismi di parte terza che effettuano le certificazioni di conformità comunitaria. In tal senso, signor Presidente, la vicenda di Viareggio diventa emblematica. Essa è imputabile al cedimento dell'asse del carro merci, prodotto nel lontano 1974 nella ex Repubblica democratica tedesca, di proprietà della società statunitense GATX Rail, con sede europea a Vienna, immatricolato presso le ferrovie tedesche Bahn; le verifiche sullo stesso sono state effettuate da Cima riparazioni di Bozzolo (Mantova), officina certificata in Germania. La proprietà ha fornito gli assi, i quali non sono stati sottoposti a verifica ad ultrasoni, in quanto né richiesto né dovuto dall'officina. In un sistema in cui vi è la presenza di una pluralità di soggetti, come evidenzia il caso in esame, è chiaro che il governo della sicurezza deve essere ripensato. Al contrario, non si è ancora provveduto in tal senso. In particolare, con riferimento al trasporto ferroviario di merci pericolose, esiste in Europa una uniforme disciplina, il cosiddetto RID, mentre il settore relativo al piano di manutenzione dei carri non è omogeneo nei Paesi UE. Ad esempio, in Italia per effettuare i controlli si usano gli ultrasuoni, mentre in Germania si usa un sistema di tipo magnetico. Senza entrare nel merito dei due sistemi, da questa diversa modalità di verifiche appare evidente la necessità di procedere ad un'analisi degli standard di sicurezza europei e della loro adeguatezza ai sistemi di controllo nazionali, ad un esame della corretta ed uniforme interpretazione delle direttive comunitarie in tutti i Paesi dell'Unione europea. È necessario, insomma, individuare "chi fa cosa" per risalire alle precise responsabilità. Ma soprattutto è indispensabile verificare la puntualità dei controlli, in quanto la più stringente normativa non produrrà alcun effetto se non accompagnata da rigorose ed effettive verifiche. Inoltre, in riferimento all'Italia appare inappropriato che le verifiche sui carri vengano fatte su base temporale e non in base al chilometraggio o alle tonnellate trasportate, che non esista un archivio informatico centralizzato sulla sulla tracciabilità del materiale circolante e, quel che è peggio, che non esistano certificazioni e qualificazioni da parte di organismi terzi indipendenti degli agenti privati che compiono le manutenzioni. E' opportuno quindi che si individui un organo pubblico, autonomo e indipendente,

l'ingegner Alberto Chiovelli, nella recente audizione alla 8a Commissione del Senato, le maggiori difficoltà consistono nel reclutamento del personale tecnico che possa assicurare una continuità con le attività sinora svolte in materia di sicurezza dalle ferrovie. Per di più lascia interdetti il fatto che la stessa Agenzia nazionale non proceda a controlli o verifiche sistematiche, ma ad un controllo dei processi. Ovvero, essa non esplica controlli sul materiale rotabile, ma verifiche meramente formali sugli operatori ferroviari per valutare la loro idoneità a gestire i processi che costituiscono la catena della sicurezza. Ovvero essa controlla i controlli! In tal senso anche l'Agenzia europea non svolge controlli, ma esplica un'attività esclusivamente di regolamentazione. Ciò pare inappropriato e non in linea a quanto opportunamente accade nel sistema europeo del trasporto aereo, cui sarebbe opportuno conformarsi. le ragioni sopra esposte, affinché non si abbia più a verificare una tragedia come quella di Viareggio, chiediamo al Governo che si adoperi subito

È inoltre necessaria la piena applicazione della Convenzione relativa al trasporto ferroviario internazionale (COTIF) per consentire la tracciabilità del materiale circolante e l'individuazione, nel possessore, del responsabile unico di tutte le fasi di vita dello stesso materiale come previsto dal Contratto di utilizzazione uniforme Ma soprattutto è necessario - signor Presidente, in conclusione - che si provveda al più presto a stanziare fondi adeguati per la messa in sicurezza del nostro sistema ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose soprattutto nei nodi urbani e nelle aree ad alta densità abitativa, e che si permetta all'organo di controllo preposto, l'Agenzia nazionale, di funzionare a pieno regime dotandosi di personale con le necessarie competenze tecniche. Non devono più esistere sciagure come quella di Viareggio non devono essere queste a farci aprire gli occhi su prassi e circostanze che in un Paese civile dovrebbero essere fuori regola già da tempo immemorabile.

È quindi importante che il dibattito che oggi si svolge in Aula abbia una concreta e rapida attuazione per gli impegni che il Governo vorrà assumersi. In un mercato che è ormai di dimensione europea e con la fine del presidio dei monopolisti, diventa indispensabile che il sistema della sicurezza sia comunitario. Moltissimi soggetti operano nei trasporti ferroviari: il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie, gli operatori del trasporto e della logistica che comperano comperano il servizio di trazione ferroviaria, società che noleggiano carri e locomotive, aziende di manutenzione ordinaria e straordinaria dei carri, industrie produttrici di materiale rotabile. È questo, indicativamente, l'elenco dei soggetti che compongono la filiera del trasporto ferroviario merci in un contesto di liberalizzazione, come quello in cui oggi ci troviamo ad operare. Un settore che per circa un secolo ha vissuto in un regime di regolazione monopolistica e che affronta in Europa il passaggio alla competizione senza un compiuto sistema di regole per la sicurezza che tenga conto in modo adeguato della frammentazione industriale, effetto indotto dal processo di liberalizzazione. Si è passati da una sicurezza di sistema, assicurata dal produttore monopolistico ed integrato del servizio, ad una sicurezza frutto dell'azione concertata di una pluralità di soggetti, senza che si sia acquisita la consapevolezza di questa radicale trasformazione di scenario. Non mancano, è vero - come altri hanno ricordato su scala nazionale le regole per la sicurezza dell'esercizio ferroviario; anzi, direi che in tutta Europa sono rigide, rigorose e capaci di assicurare uno standard complessivamente elevato di *performance* del trasporto ferroviario. Quello che però forse sinora è mancato è un processo di adattamento del modello di sicurezza al diverso contesto istituzionale del mercato ferroviario comunitario, reso più articolato e complesso dal passaggio dal monopolio alla liberalizzazione. Norme che restano rigorose nella loro formulazione originaria rischiano, in questo nuovo sistema e panorama, di essere meno efficaci perché la quantità e la qualità degli attori che partecipano al processo di erogazione del servizio è radicalmente cambiata rispetto alla situazione nella quale queste regole erano state emanate. Nel contesto dell'ambiente monopolistico, spettavano, di fatto e di diritto, i compiti di coordinamento della filiera industriale, compreso il presidio della sicurezza del sistema, al monopolista. Questo assetto è stato inevitabilmente superato, senza che le regole tenessero in sufficiente conto i costi nascenti di coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono alla erogazione del servizio e dall'altro la conseguente suddivisione delle responsabilità. Anzi, l'impressione che emerge in questo mercato ferroviario liberalizzato è che i diversi soggetti che partecipano alla filiera industriale tendano a proteggere i profili della propria responsabilità, scaricando su altre componenti del processo un compito di coordinamento di sistema. L'Europa ha ormai comunemente convenuto sull'idea che la rete debba restare nella proprietà dello Stato, mentre il mercato ferroviario che si apre alla competizione è costituito dai servizi di trasporto. Nel caso del trasporto ferroviario delle merci, che è anche il primo ad essere stato aperto alla concorrenza, oltre alla complessità del numero dei soggetti che operano, spesso in una catena sequenziale di operazioni, si è sottovalutata la dimensione del mercato del trasporto ferroviario merci. Per l'Italia, più della metà dell'intero trasporto ferroviario delle merci è traffico di *import* e/o di *export*: origina o è destinato in un territorio diverso dallo Stato nazionale. Con la liberalizzazione si è messa in discussione un'organizzazione del mercato che era basata su un regime di cooperazione tra monopolisti nazionali; sistema costituiva il modello di funzionamento nel processo di erogazione del servizio. Lo scenario della competizione è dunque cambiato ed accade che per presidiare un mercato complesso come quello europeo si determinino accordi per la fornitura di servizi di trazione tra imprese ferroviarie: l'interfaccia verso il cliente è uno solo dei soggetti produttori del servizio, che poi affida in concessione ad altre imprese ferroviarie spezzoni di tratte, per evitare di affrontare costi di investimento spesso elevati per presidiare direttamente l'intero processo di erogazione del servizio.

diventa indispensabile che il sistema di regole per la sicurezza sia di carattere comunitario: una dimensione esclusivamente nazionale ormai non è più sufficiente. La manutenzione dei carri, per esempio, storicamente determinata a tempo, rischia di non tenere conto dei livelli di sfruttamento economico del bene: parametri di sicurezza adatti ad una ferrovia storica del monopolio possono risultare non pienamente adeguati in un contesto di maggiore sfruttamento degli *asset* determinato dalle liberalizzazioni:

che voglio citare brevemente. Il primo impegno è quello rivolto ad aumentare il livello di sicurezza del trasporto ferroviario in tutta la rete nazionale, sostenendo innanzi tutto l'incremento degli investimenti economici. impegno mira a garantire la puntuale applicazione delle norme comunitarie, adottando contestualmente un sistema di controlli più incisivo ed indipendente. l'impegno a favorire la piena applicazione delle procedure COTIF (con una chiara distinzione tra la figura dell'impresa ferroviaria, dell'utilizzatore e del manutentore, stabilendo compiti e responsabilità di ciascuno) l'impegno ad adottare misure tecniche estremamente rigide per il trasporto su rotaia di merci pericolose. E ancora, un l'impegno a porre in essere ogni atto di competenza, volto a garantire una chiara tracciabilità delle attività di manutenzione dei carri, anche attraverso l'istituzione di un ente pubblico legato alla certificazione degli impianti di manutenzione dei carri medesimi; l'impegno ad agire in sede comunitaria, al fine di aggiornare le regole per la revisione dei carri e delle carrozze ferroviarie, in base a criteri che privilegino sia il dato temporale sia quello relativo al chilometraggio e al peso delle merci effettivamente trasportate; in ultimo, l'impegno a valutare l'opportunità di costruire nuove tangenziali ferroviarie destinate al trasporto merci. Questi sono gli impegni che la mozione del Gruppo dell'Italia dei Valori richiede al Governo e che ci auguriamo possano trovare il voto favorevole dell'Aula e il consenso del Governo.

Signor Presidente, signor vice ministro Castelli, onorevoli colleghi senatori, tutti purtroppo abbiamo ben presenti nella nostra memoria le immagini della tragedia di Viareggio, il più grande disastro ferroviario del nostro secolo:

Non sto a ripercorrere tutte le valutazioni dei tecnici e le immagini trasmesse dai *media* di quel primo vagone dietro il locomotore che è deragliato, trascinando le altre

agli effetti: 30.000 litri di GPL, che hanno coinvolto un'area lontana circa 400 metri dal luogo del deragliamento, hanno determinato un bollettino che nei giorni si è andato sempre più appesantendo quanto al numero dei morti,

Alcuni numeri sono già stati fatti, ma oggi mi permetto di riproporli qui, in Aula: nei primi 6 mesi del 2009 sulla rete ferroviaria italiana hanno circolato 4.394 carri con merci pericolose, dei quali 86 erano di proprietà delle Ferrovie dello Stato, 283 di privati e immatricolati in Italia, 1.834 immatricolati nel parco tedesco e 1.420 francesi; gli altri provenivano da Polonia, Austria e Svizzera. Com'è già stato detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, il carro, che era di proprietà della GATX Rail, era stato revisionato

Terminate queste premesse, considerato che i sistemi tecnologici nel campo della sicurezza sviluppati in Italia sono tra i più moderni d'Europa e sono stati anche presi a modello in diversi Paesi europei, anche se resta da completare l'installazione delle apparecchiature di sicurezza a bordo dei treni, direttive e regolamenti comunitari disciplinano le condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario in Italia, come anche nel resto d'Europa, sulla base di severe normative tecniche, per quanto attiene sia alla manutenzione sia alla circolazione dei carri ferroviari.

il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che ha assunto importanti responsabilità in alcuni campi che mi permetto di elencare: emanazione di norme e standard di sicurezza della circolazione ferroviaria; ammissione tecnica di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione; rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione della sicurezza; attività di indagine ed *audit*, nonché di monitoraggio sull'attività delle imprese ferroviarie. Personale che operava presso Rete ferroviaria italiana (RFI) è stato destinato nei settori in cui ha assunto la responsabilità l'Agenzia; attualmente però risultano scoperte posizioni di grande importanza nel sistema dei controlli che ancora sono alle dipendenze di RFI. A tal fine risulta indifferibile una loro destinazione nell'organico dell'Agenzia. L'attuale sistema del presidio della sicurezza ferroviaria in Italia, così come delineato dal decreto legislativo n. 162 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/49/CE, è fondato sulla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori della rete; la direttiva comunitaria 2008/110/CE introduce le figure di nuovi soggetti con compiti in materia di sicurezza che, nello spirito della direttiva stessa, devono portare ad un rafforzamento della sicurezza del sistema; fra tali nuovi soggetti saranno previsti la figura del detentore del carro e dell'entità di manutenzione. Ad oggi però non esiste, neanche a livello comunitario, una direttiva precisa in materia di certificazione delle officine preposte alla manutenzione e alla revisione del materiale rotabile; per questo è necessaria una riflessione sul sistema delle revisioni a tempo del materiale rotabile destinato al trasporto merci che potrebbe risultare insufficiente considerato che con la liberalizzazione l'utilizzo dei carri merci si è fatto particolarmente intensivo. Va poi ricordato e sottolineato che ad oggi non esistono regole condivise per i piani di manutenzione dei carri fra i vari Paesi europei.

2008/110/CE e 2007/58/CE che riguardano rispettivamente la sicurezza e la interoperabilità; e la interoperabilità; ad attuare, con decreto legislativo, la normativa europea (direttiva 2008/68/CE) relativa al trasporto di merci pericolose su ferro, esercitando la delega recata nella legge comunitaria per il 2008;

i soggetti che hanno il compito di rilasciare le certificazioni; le attività da compiere per verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo dei soggetti certificati.

autostrade del mare; a richiedere al gruppo Ferrovie dello Stato che vengano privilegiati gli aspetti relativi alla sicurezza della circolazione rispetto ai processi industriali e che, quindi, venga posto in essere ogni sforzo per garantire la sicurezza;

continuato a scandire i giorni che sono trascorsi da quella terribile notte, ed il nostro Gruppo ha ritenuto non solo necessario, ma urgente affrontare compiutamente qui, nell'Aula parlamentare, un dibattito chiaro dal quale risultino le responsabilità di quanto accaduto e sollecitare precise azioni concrete e coerenti che evitino che ciò si ripeta. L'incidente non è stato frutto di una causalità, ma ancora nessun responsabile è stato individuato e perseguito perché non ha fatto ciò che doveva fare. Questo primo atto è indispensabile per dare credibilità a ciò che si dichiara di voler fare per evitare che tali episodi si ripetano in futuro. Quello di Viareggio non è il solo incidente avvenuto negli ultimi mesi. Le audizioni del ministro Matteoli e del commissario Tajani hanno prodotto sino ad oggi: da parte del Ministro la promessa a riferire «in modo più concreto e dettagliato i risultati di ulteriori accertamenti» e dal secondo la notizia di «una conferenza europea a settembre» per presentare in quella sede «la proposta di un sistema europeo di controlli del settore». Ed infine l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ingegner Moretti, dichiara che i certificati di sicurezza vengono rilasciati da FS attraverso una struttura interna a Rete ferroviaria italiana. E nel mentre afferma che auspica un'autorità per la sicurezza interna alle ferrovie, l'unica vera proposta è il macchinista unico per non avere più bilanci in rosso a causa della sicurezza. La confusione di intenti e la babele di linguaggi mi paiono l'unica cosa certa in questo momento. La preoccupazione non è solo dettata dal fatto che il Governo del "fare" adesso lo possiamo declinare con il Governo del "fare... confusione", ma preoccupa che nel contempo i treni continuino a viaggiare, compresi quelli che trasportano sostanze pericolose, e cioè le famose bombe a cielo aperto, su vagoni che non sono stati sottoposti ad una fermata per un controllo intensivo di verifiche e di manutenzione straordinaria. Insomma nulla, solo parole... parole, parole. In questi mesi abbiamo ripetutamente sollecitato il Governo e l'azienda ad intraprendere con decisione un processo dì modernizzazione del nostro sistema ferroviario, fatto di adeguamenti legislativi, di recepimento di normative europee che consentano di inserirci in modo adeguato nella futura liberalizzazione del mercato ferroviario, di investimenti infrastrutturali e potenziamento delle risorse umane in grado di affrontare il futuro delle ferrovie e non solo di utilizzare al meglio ciò che ci consegna il passato. Abbiamo proposto ripetutamente, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza ferroviaria, di rendere pienamente operativa l'Agenzia italiana per la sicurezza delle ferrovie, dotandola di mezzi e personale in grado di svolgere pienamente le funzioni a cui è preposta. In attesa di tutto ciò si doveva, e si poteva fare di più. E per la pericolosità delle merci e delle situazioni operative che coinvolgono il nostro sistema ferroviario si deve e si può fare di più. La gestione della rete, intanto. Non bastano solo le tecnologie legate al controllo della segnaletica e dell'incanalamento dei flussi, ma il passaggio da un mercato monopolistico ad un mercato liberalizzato necessita di tempi e modalità di accompagnamento che non esimono il Gruppo Ferrovie dello Stato dal comportarsi come soggetto pubblico. Infatti, ancorché società per azioni, Ferrovie usufruisce di cospicui finanziamenti statali nell'infrastrutturazione, nell'acquisto di mezzi ed in tutte le scelte gestionali. In una recente audizione in 8a Commissione, l'ingegner Moretti, ad una precisa domanda ha risposto che il nostro sistema ferroviario di trasporto merci è in grado di affrontare un consistente incremento di questa modalità di trasporto in quanto lavora al di sotto delle proprie potenzialità. Per accompagnare tutte le scelte necessarie ad incrementare questo obiettivo è necessario, però, partire innanzitutto dalla riprogrammazione infrastrutturale della rete e dei nodi quali le stazioni terminali, i raccordi, i porti e gli interporti, che individui la creazione di corridoi e nodi espressamente dedicati alle merci e che non si sovrappongano al trasporto passeggeri; evitando così di far transitare, soprattutto le merci pericolose,

dove un incidente, sempre possibile nelle attività umane, può avere gli effetti di una strage come avvenuto appunto a Viareggio.

Ho letto con attenzione tutte le mozioni presentate: rispondono pressoché tutte alla medesima esigenza, cioè quella di allertare le autorità competenti, per la via del Ministero competente, a fare in modo che vengano rimosse le cause strutturali che determinano

determinare e circoscrivere le responsabilità, non tanto per il desiderio di punire, quanto per il desiderio di dare esempio a chi è preposto alla funzione di vigilanza e controllo

dopo i drammatici eventi di Viareggio della notte tra il 29 ed il 30 giugno, mentre la lista delle vittime continua a crescere, dopo decine di feriti in gravissime condizioni e milioni di euro di danni, ci troviamo finalmente a discutere di sicurezza nel trasporto ferroviario. Come ha ricordato il senatore D'Alia, è una sciagurata abitudine quella che ci induce a discutere di rischi e sicurezza solo dopo che sono accaduti fatti drammatici: è una prassi che dovremmo impegnarci tutti, almeno per quanto possibile, a superare. È una regola - quella di discutere dopo - che oggi applichiamo al trasporto ferroviario, ma è valsa per il rischio sismico, per la sicurezza nel lavoro, continua a valere per la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente o per i rischi collegati ai mutamenti climatici. Prima di entrare nel merito delle mozioni, permettetemi da fare alcune brevissime considerazioni. Noi viviamo in una società tecnologica segnata dalla complessità e dalla quantità. È sempre più difficoltoso controllare i sistemi che la contraddistinguono e la quantità enorme di mezzi, merci, materiali ed informazioni che la alimentano. Tali sistemi complessi interagiscono con l'ambiente e cambiano la vita, giorno dopo giorno, di miliardi di persone: producono opportunità, aiutano ad elargire servizi di ogni genere, ma generano anche nuovi rischi sempre più difficili da prevedere e contenere. Dobbiamo allora iniziare a considerare questi rischi, sul lavoro, nei trasporti, nella produzione e nell'ambiente, in modo diverso dal passato, sia per garantire una corretta prevenzione (cioè maggiore sicurezza per tutti) sia per le conseguenze che possono provocare in tutti i campi: da quello umano a quello economico ed ambientale. In questo contesto, la sicurezza - innanzi tutto, quella per gli esseri umani è destinata a diventare qualcosa di molto diverso dal passato, qualcosa di dinamico, di adeguato ad una società che muta giorno dopo giorno. La sicurezza non può essere ridotta ad un dato statistico; ha bisogno di competenze e di un lavoro ampio ed articolato, che sappia porre al centro la vita degli uomini e delle donne che vivono nelle città, che producono, che viaggiano, che consumano. Come richiamano tutte le mozioni, è urgente superare un grave ritardo e dare corso al rapido decollo dell'Agenzia italiana per la sicurezza delle ferrovie. Occorre dotarla di risorse umane, di adeguate competenze, dei mezzi tecnici e finanziari necessari alla sua funzionalità. Il Governo deve ancora emanare gli appositi decreti: può essere l'occasione per sperimentare, pur a partire dallo specifico oggetto della discussione e nei limiti del decreto legislativo n. 334 del 1999, una visione più ampia della sicurezza. Proprio perché la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti non può più essere rinchiusa nell'ambito nazionale, occorre dare immediato seguito alla ratifica e stipula di tutti gli accordi in essere ed ai quali fanno riferimento le mozioni, fare propri gli standard europei, con la consapevolezza che tali accordi, ovunque siano assunti, non potranno più aver una valenza perpetua ma dovranno essere periodicamente rivalutati e rielaborati, in un'ottica integrata di competenze e di dinamica attenzione all'evolversi della qualità e quantità dei rischi. Particolarmente importante, poi, è affrontare la questione della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, aprendo il capitolo della progressiva esclusione del loro transito dai centri urbani. Questioni come la costruzione di nuove cinture ferroviarie e di comunicazione, che tendono ad escludere le città dal rischio derivante dal transito delle merci pericolose, l'attuazione di adeguati protocolli di certificazione di sicurezza, un'attenta regia di un'agenzia che non sia un nuovo carrozzone ma uno strumento efficace di studio, analisi, intervento

dagli stessi operatori del settore - non può essere ridotta ad una mera questione economica o ad un'astratta valutazione sul rapporto tra lavoro umano e automazione degli impianti e dei controlli. Il metro di giudizio deve essere quello della prudenza e della sicurezza. Ricordo che a Viareggio è stato proprio l'intervento del capostazione ad evitare che un incidente gravissimo si trasformasse in una vera e propria immane catastrofe. Occorre che queste mozioni non rimangano lettera morta o atti formali dovuti e scaturiti a

poiché non è nelle nostre possibilità azzerare ogni forma di rischio, bisogna avere presente che gli incidenti possono purtroppo accadere. Dunque, prevenzione, controllo ma anche assistenza. L'assistenza alle vittime, a chi ha avuto danni materiali e morali è uno dei capitoli integranti della questione sicurezza. Partendo dai fatti di Viareggio, voglio richiamare due aspetti che mi sembrano centrali. La ricostruzione delle responsabilità coinvolte ha portato all'individuazione di una pluralità di soggetti, rendendo l'*iter* dei risarcimenti pericolosamente complesso.

è dato dal fatto che poiché non è pensabile un arretramento in termini di liberalizzazione ferroviaria, deve essere più forte il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea, nel senso che deve essere più stretto il legame tra l'Agenzia europea e quelle nazionali. Deve esserci un controllo operato direttamente dall'Agenzia europea, in analogia a quello che accade, per esempio, nel sistema aereo, ovviamente *mutatis mutandis* essendo completamente diversi i vettori aerei da quelli ferroviari e naturalmente diversi i gradi di

della necessità di garantire un trasporto sicuro. Questo vale tanto più - e questo è il secondo elemento elemento - se parliamo di merci pericolose. Abbiamo vissuto incidenti stradali molto gravi per effetto di merci infiammabili, esplodenti e quant'altro abbiamo auspicato, a valle degli stessi, un maggior utilizzo del trasporto ferroviario per quel tipo di merci. giusto questo orientamento, ma dobbiamo imparare una lezione importantissima dai fatti avvenuti: se quello che è accaduto fosse accaduto in una galleria lunga, con altri treni in transito, oggi parleremmo di migliaia di morti

Queste semplici scelte potrebbero costituire già un forte incremento della sicurezza. Un ultimo punto riguarda l'intervento della collega che mi ha preceduto e concerne il tema assicurativo. Nel sistema della liberalizzazione, proprio perché gli attori si moltiplicano, è estremamente complessa la ricostruzione della responsabilità, ma chi ha subito danni non può aspettare i tempi lunghi dell'accertamento della giustizia. È giusto che il Governo promuova iniziative atte ad attenuare il disagio di chi ha avuto danni

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la mozione che abbiamo presentato e il dibattito di oggi vogliamo porre all'attenzione di tutto il Senato i risultati conseguiti dal vertice de L'Aquila, che sono il frutto di un lavoro lungo e paziente e pongono le basi di un ambizioso programma di riforme e di interventi, che dovrà e potrà vedere il Parlamento italiano come protagonista. La Commissione affari esteri, che ho l'onore di presiedere, insieme alla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ha avviato da tempo un'indagine conoscitiva sulla Presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale: in quella sede, abbiamo avuto modo, nel confronto diretto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia, con lo *sherpa* del Governo italiano e con i rappresentanti di enti di ricerca, di seguire la preparazione del vertice e approfondire i principali temi che ne hanno caratterizzato l'agenda. Non ci stupiamo, dunque, del successo di un evento che è stato accuratamente preparato, con una professionalità di cui dobbiamo dare atto al Governo e in particolare ai funzionari a vario titolo coinvolti. Permettetemi qui di cogliere l'occasione per dare il dovuto riconoscimento alla professionalità della nostra diplomazia, alla cui preziosa attività spero vorremo destinare, con la prossima manovra finanziaria, le risorse indispensabili a garantire quell'alto livello di professionalità e di esperienza che permetta all'Italia di svolgere un ruolo efficace e apprezzato sulla scena internazionale. In un momento di grave difficoltà per le nostre economie e per le nostre società, il vertice ha costituito un'occasione preziosa, che non è andata persa, per riaffermare la necessità di una efficace *governance* mondiale. Come ha detto bene il Capo dello Stato a L'Aquila, le crisi che stiamo vivendo da un anno sono «La prova inconfutabile che è con un mondo globale che dobbiamo fare i conti, che è un mondo globale quello che si deve governare. Nessun Paese e nessun Continente può fare da solo». Questa consapevolezza ha animato e indirizzato i lavori della Presidenza italiana, che ha voluto avviare, proprio con il G8 de L'Aquila, la costruzione di una nuova architettura della *governance* mondiale, coinvolgendo le grandi economie emergenti. Non esiste ancora un consenso sulla forma e la composizione futura di un G8 riformato; l'Italia ha quindi efficacemente adottato diversi formati, puntando sul valore aggiunto di ciascuno. Si sono svolti a L'Aquila: una sessione del solo G8; del G8 allargato a Brasile, Cina, India, Messico, Sud Africa ed Egitto; un Forum delle maggiori economie per affrontare i problemi dell'energia e del cambiamento climatico; una sessione del G8 con i *partner* africani per discutere l'impatto della crisi economica sui paesi in via di sviluppo; infine, una sessione sulla sicurezza alimentare con tutti i *leader* presenti al vertice. Il gruppo dei Paesi che costituiscono il G8, per la comunanza dei valori cui essi si ispirano, continua a svolgere un prezioso ruolo di stimolo e di indirizzo per una *governance* mondiale che tuttavia va resa più articolata e rappresentativa, come proprio a L'Aquila, con successo, si è iniziato a fare. Ed è stata questa articolazione più rappresentativa della complessa realtà mondiale che ha permesso al vertice di conseguire risultati significativi e assumere impegni ambiziosi la cui attuazione e sviluppo dovremo seguire con particolare attenzione nel prossimo futuro. Il primo risultato consiste nella decisione di chiudere entro il 2010 i negoziati di Doha sulla riduzione delle barriere agli scambi internazionali. Mai come in questo momento occorre infatti dare una risposta chiara alle tensioni protezionistiche che agitano la scena politica di tanti Paesi. Lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale, la stessa crescita dei Paesi più poveri, necessitano un più elevato tasso di liberalizzazione dei commerci. E proprio verso i Paesi poveri il vertice ha voluto ribadire impegni di aiuto e varare programmi più efficaci e ambiziosi di quanto previsto in passato. Faccio qui riferimento al programma di sicurezza alimentare, per il quale si è prevista una dotazione finanziaria di 20 miliardi di dollari. Innovando rispetto al passato, il programma mira ad accrescere le potenzialità delle produzioni agricole dei Paesi poveri. L'esperienza mostra come politiche limitate al semplice aiuto alimentare, se risolvono le esigenze più pressanti delle popolazioni, non incidono sui problemi strutturali, anzi hanno generato in alcuni casi effetti perversi. Da ciò l'impegno a fornire assistenza tecnica, a formare le popolazioni rurali, per garantire una mutazione della loro reale capacità di produzione. Sono questi Paesi che dobbiamo responsabilizzare di più, migliorando le strutture amministrative e le capacità di governo. In fondo, è questo il messaggio portato al continente africano dal presidente Obama, che si è rivolto ai *leader* degli Stati africani richiamandoli alle loro responsabilità. Un mondo, dunque, più rispettoso di regole e comportamenti politici fondati sulla responsabilità. L'adozione di nuove, più efficaci regole e metodi di supervisione per ristabilire fiducia nei mercati finanziari e prevenire che altre crisi si producano in futuro, è stato un altro degli obiettivi perseguiti dal G8. Queste regole sono state cristallizzate nel cosiddetto "Lecce Framework", una serie di principi promossi dalla Presidenza italiana - e in particolare dal nostro Ministro dell'economia per sviluppare standard comuni nell'economia e nella finanza mondiale, volti a garantire la correttezza, l'integrità e la trasparenza delle relazioni finanziarie. Si è stabilito, inoltre, di potenziare la cooperazione internazionale per combattere la corruzione, il riciclaggio del denaro, il terrorismo finanziario e l'evasione fiscale attraverso l'attuazione di regole comuni internazionali rafforzate, sostenendo le iniziative nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Il richiamo ad una dimensione etica nei rapporti economici e finanziari è stato formulato con forza, proprio in questi giorni, nell'ultima enciclica di Papa Benedetto XVI, un richiamo al profondo valore dell'economia sociale di mercato da parte di un uomo come ha giustamente notato un nostro autorevole collega - che unisce all'autorità spirituale il suo essere cittadino di un Paese che affrontò e vinse la sfida della ricostruzione, con Konrad Adenauer e Ludwig Erhard, proprio ricorrendo all'economia sociale di mercato. L'attenzione ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile ha condotto il dibattito in seno al G8 a concentrarsi su un altro grande dossier: quello relativo al cambiamento climatico e, conseguentemente, alle nuove sfide per le politiche energetiche. Questo dibattito si è svolto con il pieno coinvolgimento delle principali economie emergenti e si è concluso con una presa di posizione comune che reca l'impegno su un ambizioso programma di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e pone le basi per un accordo globale alla Conferenza di Copenaghen del prossimo dicembre 2009. Le grandi economie hanno convenuto di impegnarsi per impedire l'aumento della temperatura media del pianeta soprattutto per uno sforzo comune nello sviluppo della ricerca, nelle energie alternative, nelle politiche di risparmio energetico. Dietro questo impegno vi è l'ambiziosa sfida di una profonda trasformazione tecnologica di cui l'Italia può e deve essere protagonista. con il più grande interesse che si guarda all'attività oltre oceano della nostra principale azienda automobilistica, alla sfida che la vedrà protagonista in un cambiamento di stili di vita e di consumi, cui la nuova Presidenza statunitense ha impresso uno straordinario salto di qualità. Vediamo così, colleghi, quanto le scelte de L'Aquila non siano lontane dalla nostra vita, ma influenzino in modo diretto le prospettive delle nostre società e debbano segnare anche la nostra attività di legislatori. A L'Aquila i *leader* del pianeta si sono poi concentrati sui principali temi politici dell'Agenda internazionale. Ne è uscito innanzi tutto un impegno forte per la riuscita della Conferenza del riesame del Trattato di non proliferazione nucleare che si terrà il prossimo anno, nella prospettiva condivisa, mai formulata con tanta chiarezza in un documento del G8, di «un mondo senza armi nucleari». La minaccia nucleare è una delle grandi sfide cui la comunità internazionale si trova di fronte. È un impegno che ci è costato e ci costa anche sacrifici. In occasione del G8 dei Ministri degli esteri di Trieste è stata approvata una strategia di stabilizzazione dell'Afghanistan. Nei prossimi giorni ci troveremo a discutere in Senato del provvedimento sul rinnovo della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Il nostro rinnovato e rafforzato impegno in Afghanistan è il prodotto di scelte che abbiamo assunto insieme agli altri *partner* proprio in occasione del vertice del G8. È un impegno per la pace e la stabilità al quale dobbiamo restare coerenti perché il sacrificio dei nostri soldati, da ultimo di Alessandro Di Lisio, al quale rivolgo un pensiero commosso, non sia inutile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il vertice de L'Aquila ha proposto questioni e temi sui quali saremo chiamati a riflettere; fra questi, le misure da intraprendere per garantire il rilancio della nostra economia. Lo abbiamo voluto dire con chiarezza nel dispositivo della nostra mozione. Occorre dare un puntuale seguito agli impegni relativi al riassetto del sistema di regolazione del mercato finanziario e occorre soprattutto che l'Italia si impegni adottando le necessarie riforme strutturali al fine di garantire che la ripresa economica si fondi su più solide e sostenibili basi. La crisi deve essere un'occasione per ristrutturare e rendere più competitiva e forte la nostra economia. È questa la sfida che abbiamo di fronte; sono questi gli impegni che le conclusioni del G8

infatti, che il merito sia ascrivibile certamente al Governo e al Presidente del Consiglio; certamente al ruolo fondamentale ed insostituibile del nostro Capo dello Stato; certamente a

che funge spesso da contraltare alla effettiva concretezza operativa degli stessi nell'offrire risposte adeguate ai problemi del mondo, i risultati raggiunti durante l'ultimo incontro tra i *leader* a L'Aquila sono condivisibili e sostanzialmente accettabili, eccezion fatta per alcuni impegni presi dal Governo italiano, a nostro avviso di poca sostanza anche rispetto agli stessi impegni presi dagli altri Paesi. Come si potrebbe definire altrimenti, nell'ambito dell'ammontare di 20 miliardi di dollari di aiuti complessivi previsti per l'Africa, il contributo del nostro Paese di soli 450 milioni di dollari, fanalino di coda per intensità d'aiuto rispetto a tutti gli altri Paesi Paesi partecipanti? A maggior ragione, se si considera che negli ultimi anni, come anche sottolineato dalle associazioni a sostegno dell'Africa, l'Italia ha disatteso i precedenti impegni presi, riducendo drasticamente l'ammontare di risorse finanziarie previste a sostegno del continente africano. Rileviamo, dandone atto al Governo, come lo stesso si sia fatto promotore di soluzioni e proposte sulla crisi finanziaria internazionale; ma con la stessa obiettività notiamo come il riscontro pratico della buona volontà, anche con gli interventi nazionali posti in essere a sostegno del sistema economico italiano contro la crisi, sia stato poco concreto e poco focalizzato sulle necessità reali degli operatori economici e, innanzi tutto, sui temi che riguardano la famiglia. Pur accogliendo con piacere il palese tentativo di pianificare una serie di misure di carattere fiscale a sostegno delle imprese, peraltro confermato nell'ultimo decreto anticrisi in discussione alla Camera, molto poco si è fatto per sostenere i primi attori del sistema economico, cioè le famiglie italiane. L'unico vero modo di proteggere le stesse dai dirompenti effetti della crisi - noi lo diciamo da tempo - è prevedere l'introduzione del quoziente familiare all'interno dell'ordinamento tributario italiano (una delle riforme strutturali cui si faceva cenno prima) e dispiace che la maggioranza, pur avendolo inserito tra i proclami elettorali, lo abbia messo troppo in fretta nel dimenticatoio. Il baricentro delle misure a sostegno della crisi sembra essere fin troppo spostato in favore delle imprese. E questo, sia chiaro, non è un male. Lo potrebbe diventare però nella misura in cui i pur apprezzabili interventi siano fin troppo rivolti verso la previsione di incentivi fiscali. Il vero problema delle aziende, oggi, è infatti la mancanza di risorse finanziarie liquide per far ripartire gli investimenti, casi migliori, e per impedire stati di insolvenza già in stato terminale, nei casi peggiori. Dunque notiamo quanto poco sia stato fatto per incentivare realmente le banche ad impedire "l'asfissia finanziaria delle piccole e medie imprese italiane",

e crescente occupazione nel mondo. Preoccupazione che, purtroppo, non è sfociata in misure concrete a favore dell'occupazione stessa, che è il perno fondamentale dello stato di salute dei cittadini e delle famiglie, come lo stesso Santo Padre, nell'offrire sostegno a quanti soffrono il dramma della disoccupazione, ha sottolineato nel recente Angelus, dicendo che: «solo restando fedeli ai valori della famiglia e del rispetto della vita umana, della giustizia sociale e con la disponibilità alla fatica e al sacrificio, si può costruire una società solidale e fraterna». In occasione dell'incontro dei *leader* mondiali, inoltre, molto ci si aspettava sugli impegni e sulle proposte da prendere sui temi ambientali ed energetici. Le aspettative - notiamo con piacere - hanno trovato risposta negli impegni presi circa la riduzione delle emissioni globali di gas serra di almeno il 50 entro il 2050 e la promessa di contenere l'aumento medio delle temperature globali entro i 2 gradi centigradi. Dispiace che non abbiano preso parte formalmente agli impegni Paesi a forte emissione di anidride carbonica come la Cina e l'India. Molto poco si è stabilito in tema di risposte all'emergenza idrica e della salute, soprattutto per i Paesi a maggior concentrazione di povertà e malattia come l'Africa. Per quest'ultimo aspetto proponiamo che l'Italia assuma sempre più i panni di *partner* privilegiato, vista anche la sua vicinanza con i Paesi a Sud del Mediterraneo. In tema di impegni a sostegno del settore energetico e dell'ambiente restiamo in attesa di capire come il Governo intenda dare concretezza ai citati impegni presi. Se accogliamo con estremo piacere la volontà e l'impegno preso a prevedere il ritorno del nucleare nel nostro Paese, scopriamo con stupore come, prendendo spunto da una recente ricerca, l'Italia, storicamente ai livelli più bassi d'Europa in fatto di investimenti destinati alla ricerca in generale, nel settore energetico, dopo la Francia, presenti il più elevato investimento *pro capite* (6 euro contro i 5,2 della Germania, i 2,8 della Gran Bretagna, gli 1,9 della Spagna). Circa il 30 per cento degli investimenti sono destinati al nucleare (ultimo dato 2005, ma la situazione non sembra essere cambiata), il 14 alle rinnovabili, il 10 all'efficienza, il 7 all'idrogeno, il 25 alle altre tecnologie. Nonostante questa evidente base di eccellenza, il sistema Italia non è emerso in questi anni come luogo di produzione dell'innovazione in campo energetico, in quanto gli investimenti non si sono tradotti in brevetti ed hanno sofferto di dispersione e poca concentrazione degli interventi. Dunque, potenzialmente, il nostro Paese potrebbe essere all'avanguardia in campo energetico, ma siamo costretti ancora, e da anni, a pagare le bollette molto più dei nostri colleghi europei. Le stesse fonti rinnovabili non riusciranno mai a svilupparsi in modo concreto se non si snelliscono ed uniformano le procedure di autorizzazione, non si limitano i troppi veti locali, in definitiva la politica energetica non torna ad essere appannaggio, competenza e prerogativa esclusive dello Stato.

tema particolarmente delicato e complesso che verosimilmente non si riesce ad esaurire nella funzione e nel ruolo, anche decisorio, che possono avere i G8, in versione più o meno allargata, e che implica una discussione sulla riforma dei modelli organizzativi e decisionali internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite, di cui il G8 non può essere un debole surrogato. Si pone anche il tema, però, di una maggiore responsabilizzazione della nostra attività di politica economica, finanziaria e di *welfare* interno, che ha bisogno di quelle riforme strutturali, senza le quali la ripresa sarà per noi un problema e non una risorsa ed un valore raggiunto. Per questo anche nella nostra mozione abbiamo ripreso questi temi, a cominciare da quello della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, per passare al tema della riforma del sistema previdenziale e del sistema del *welfare*

è una crisi internazionale. Per queste ragioni riteniamo, pur essendo aperti ad un confronto che speriamo si possa avere in Aula anche con i colleghi di maggioranza e opposizione per vedere se è possibile su alcuni punti arrivare ad un testo condiviso, che in questa mozione si sia concentrata la morale del G8.

devono essere rispettati. Per essere noi credibili dobbiamo anzitutto essere nelle condizioni, nel nostro Paese, di applicare quelle politiche, di essere coerenti con esse e di avere la forza di adottare misure che possono essere anche impopolari, ma che certamente nel medio e nel lungo periodo costituiranno

Signor Presidente, il recente *Summit* degli 8 Grandi, che si è concluso a L'Aquila, ha formalizzato una serie di impegni che riteniamo tutti importantissimi: dalla dichiarazione sul futuro sostenibile alla dichiarazione sulla non proliferazione nucleare, contro il terrorismo, sull'energia e sul clima, sulla sicurezza alimentare. insomma un impegno a largo spettro. Vorremmo, però, soffermarci sulla tematica della crescita equilibrata e sostenibile. In sostanza, a L'Aquila si è espressa la volontà di rinnovare l'impegno globale degli 8 Paesi nei confronti dei Paesi poveri ed in particolar modo si è fissata l'attenzione sull'Africa. Si sono in sostanza prese delle misure tese a mitigare l'impatto della crisi proprio su quei Paesi in via di sviluppo che avrebbero accusato maggiormente anche anche la minor capacità nostra di intervenire. Siamo perfettamente d'accordo e completamente in linea con queste dichiarazioni. Ciò che diciamo è che bisognerebbe adesso

compiuto salti o avuto dei risultati, almeno quelli che si speravano. Pensiamo, per esempio, al fallimento delle politiche dell'accoglienza *tout

realizzate fino agli anni '90, dove la politica per la cooperazione e lo sviluppo sembrava più una lottizzazione, una spartizione geografica del globo: i socialisti avevano lottizzato l'Africa; l'Asia era appannaggio dell'allora PCI; l'America latina era terreno operativo per la Democrazia cristiana. aiuti servivano più per affermare l'influenza di queste organizzazioni e di questi partiti che non per la risoluzione dei problemi delle popolazioni di quei siti bisognosi.

regole fondanti, «possano scaturire decisioni ed orientamenti utili al vero progresso di tutti i popoli, e in special modo di quelli più poveri»;

ci si limita sostanzialmente a stanziare dei fondi per poi consegnarli alle organizzazioni più variegate, che attuano interventi isolati o comunque disorganici, o peggio ad affidare queste risorse a dei Governi tante volte corrotti che non hanno mai considerato i diritti effettivi dei loro popoli.

Quel che diciamo con questa mozione è che vanno cambiate radicalmente le politiche di aiuto a tali Paesi. Dovremmo passare dal donare esclusivamente cibo - quello che avviene oggi - ad un coinvolgimento della persona, dell'uomo nel cammino autonomo che dovrebbe fare compiere verso il benessere, i diritti e la libertà. Non dovremmo più riproporre gli errori che abbiamo visto. Non dovremmo più ingenerare quei falsi miti, quei falsi paradisi che hanno portato interi popoli ad abbandonare i loro Paesi di origine: invece che partecipare alla loro evoluzione, sono scappati verso le nostre terre promesse, che per lo più si sono rilevate fonti di dolore, sofferenza emarginazione e, a volte, anche di morte. Il nostro impegno è pertanto indirizzato innanzi tutto ad aiutare tutti i popoli del mondo a migliorare le condizioni dei propri Paesi d'origine, a credere nel loro sviluppo ed a lottare per questo, chiaramente con l'aiuto di tutta la comunità internazionale. ragione la nostra mozione chiede al Governo di orientare le proprie politiche di cooperazione, accoglimento ed immigrazione come elementi di un'unica visione che ponga al centro l'idea di dare a tutti gli uomini l'opportunità di vivere con dignità nei propri Paesi, senza essere costretti o indotti a lasciare i Paesi natii, al prezzo - come abbiamo visto - di enormi sofferenze. Inoltre, chiediamo un nuovo tipo di rapporti tra Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo, dove nei primi non continui a prevalere la ricerca e lo sfruttamento delle risorse e nei secondi venga garantito che gli aiuti siano destinati effettivamente alle popolazioni bisognose. In ultimo, chiediamo che la cooperazione allo sviluppo sia un elemento integrante della politica estera e pertanto venga indirizzata prioritariamente a quei Paesi con i quali si sono instaurati rapporti di amicizia e reciproca intesa. Abbiamo dovuto dire "prioritariamente" non potevamo chiaramente dire "esclusivamente", ma è facile anche capire che è molto più opportuno e più semplice aiutare efficacemente i Paesi con cui si hanno rapporti molteplici, che pertanto portano a conoscerne meglio meglio i bisogni e ad adottare le migliori strategie per sollevarli dal bisogno. In sostanza, la nostra mozione potrebbe essere inquadrata con una sintesi: dare ad ogni uomo l'opportunità di vivere dignitosamente nel proprio Paese.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, forse è presto per predisporre un bilancio degli obiettivi raggiunti e non raggiunti dal recente vertice G8. Possiamo però dire che, al di là delle valutazioni finali che verranno predisposte, il G8 si è svolto nel nostro Paese in una condizione di ottima agibilità politica.

a quello delle settimane precedenti, e quindi una sorta di nuova solidarietà nazionale ha permesso di trascorrere quei giorni

Noi, con la mozione che mi accingo ad illustrare, abbiamo voluto sottolineare l'importanza strategica che un incontro tra i cosiddetti grandi della terra può assumere nello scacchiere mondiale. La crescita deve essere declinata all'insegna della giustizia sociale e deve potersi sviluppare restringendo la forbice economica, cioè limitando il più possibile il divario tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri,

da queste inclusioni, anzi le chiamiamo diversamente perché riteniamo che non vi debba essere alcun fattore dominante rispetto ad un soggetto presuntivamente debole. Nella nostra mozione, però, abbiamo parlato anche dell'organizzazione del G8. In buona sostanza ancora ci chiediamo - e lo chiediamo al Governo tramite questa mozione - quali siano stati effettivamente i motivi per i quali, subito dopo il triste episodio del terremoto in Abruzzo, il Capo del Governo ha deciso di cancellare la sede de La Maddalena e di spostare il G8 a L'Aquila. È stato detto che il motivo risiedeva nella necessità di mostrare - sempre ai cosiddetti grandi della terra - il dolore della popolazione abruzzese, i danni provocati da quella immane sciagura. Si è parlato, in

La Maddalena è stata inopinatamente abbandonata; a La Maddalena sono state realizzate opere con i soldi dei sardi; a La Maddalena è stato chiesto uno sforzo organizzativo che ha comportato anche una notevole assunzione di di responsabilità nei confronti dei fornitori. Tutto ciò ha determinato debiti, ha determinato il famoso danno emergente e l'altrettanto famoso lucro cessante. Noi, con questa mozione, chiediamo che almeno ciò che è stato realizzato diventi in qualche modo patrimonio morale del nostro Paese, in maniera tale che le opere realizzate con i soldi dei sardi i soldi dei sardi possano costituire oggetto di attenzione da parte di un Governo che nel futuro dovrà sviluppare altre iniziative di carattere internazionale, che

il palazzo della «Main Conference» e tutti gli altri edifici predisposti per il lavoro delle delegazioni, nonché gli interventi di riqualificazione dell'ex Arsenale possano diventare oggetto di una manutenzione operativa, e comunque possano essere utilizzati in incontri e congressi internazionali. In buona sostanza, chiediamo che l'isola sia considerata dal Governo il luogo deputato ad accogliere nel futuro tutti gli appuntamenti che abbiano questa caratteristica. Signor Presidente, quando il Governo Prodi scelse La Maddalena, il Presidente del Consiglio e lo stesso Presidente della Regione dell'epoca dissero che quella scelta era stata informata dal desiderio di risarcire La Maddalena per ciò che in almeno 30 anni aveva dato alla politica internazionale e alla politica mondiale. Non dimentichiamo, signor Presidente, che a La Maddalena non c'era una base NATO: c'era una base americana. Non dimentichiamo che per 30 anni a La Maddalena si è convissuto con i missili a testata nucleare. Non dimentichiamo che nel giardino di casa avevamo una santabarbara che avrebbe potuto far saltare in aria tutta l'isola della Sardegna. se quello era un risarcimento, se non c'era malevolenza nelle intenzioni del Presidente del Consiglio, se quello spostamento moralmente può essere stato in qualche modo subito dal Presidente del Consiglio e dal Governo, ebbene si approvi la nostra mozione: approvando la nostra mozione, concretamente e non soltanto con formali manifestazioni di principio potrà essere restituito il maltolto.

onorevole sottosegretario Scotti, i contenuti e i temi discussi al G8 de L'Aquila, come l'economia, la finanza, i diritti umani, l'acqua e la sicurezza alimentare, obbligano ad aprire un dibattito a tutto campo nelle sedi parlamentari, soprattutto se guardiamo ai limiti e ai silenzi contenuti nel Documento di l'interdipendenza tra le economie e la crisi economica e morale che ha investito i Paesi ricchi hanno trasformato la natura del dibattito sul risanamento delle nostre economie, non più monadi di un mondo privilegiato, ma sottoposte a tutte le ripercussioni che viviamo individualmente e quotidianamente. Sbloccare un vero e proprio intreccio perverso in cui si è venuta a trovare l'economia italiana, dopo aver accumulato un ritardo di crescita che ha accentuato sia l'instabilità macroeconomica che il disagio sociale, è il nostro imperativo. Tuttavia, la risalita del debito configura una condizione insostenibile dei conti pubblici, ci espone alle pressioni del mercato internazionale e ci pone in difetto rispetto alle regole europee. Nello stesso tempo, crescita pressoché zero, inefficienza e distorsioni del sistema tributario, scarsa efficacia della politica di bilancio a finalità redistributiva contribuiscono a peggiorare gli indicatori di disuguaglianza e povertà. A frenare ulteriormente lo sviluppo economico e il tasso di crescita potenziale concorrono, inoltre, l'insufficienza dei meccanismi premianti la qualità, un contesto generale poco favorevole all'impresa ed agli utenti consumatori, l'ampiezza di settori protetti e privi di concorrenza. La politica economica è così chiamata ad agire contemporaneamente su tre fronti: sviluppo, risanamento ed equità. Contemporaneamente, perché sono inscindibili. La crescita è indispensabile per generare le risorse necessarie ad un aumento del benessere, alla riduzione della povertà, al risanamento dei conti pubblici; l'equità esige che si ponga fine a fenomeni inaccettabili di evasione ed elusione fiscale, che generano situazioni di sofferenza finanziaria che colpiscono soprattutto gli strati deboli, oltre che le generazioni future. In un regime democratico una maggiore equità è condizione indispensabile nel processo di risanamento finanziario e di rilancio della crescita. Ma c'è un quarto fronte inscindibile dagli altri tre, sul quale bisogna operare contemporaneamente: la crisi globale, il crollo delle regole che hanno tenuto in piedi le economie dei Paesi più forti e la disperata pressione di una parte maggioritaria del mondo impongono la politica della cooperazione allo sviluppo al primo piano nella ribalta internazionale. È quanto ha fatto l'Unione europea nel momento in cui, a seguito della modifica del Patto di stabilità, dichiara di riservare particolare attenzione, ai fini della determinazione del deficit, agli "sforzi di bilancio intesi ad aumentare o mantenere i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale". Stupisce che ci sia ancora la necessità di ripetere che non esiste possibilità di rilancio effettivo e duraturo delle economie occidentali se più di due terzi della popolazione del pianeta lottano lottano per sopravvivere alla fame, alla sete, alle malattie e alle guerre, che spesso hanno come concausa il cambiamento climatico. Questa visione del futuro era chiara al precedente Governo. Infatti, stigmatizzando il ritardo dell'Italia già nel 2006 rispetto agli impegni assunti internazionalmente (con un rapporto tra aiuti per lo sviluppo e PIL pari solo allo 0,20 per cento contro lo 0,33 per cento la legge finanziaria 2007, pur nella difficile situazione finanziaria del Paese, aveva marcato una significativa inversione di tendenza, con un notevole incremento degli stanziamenti per gli aiuti allo sviluppo. I fondi del bilancio del Ministero degli affari esteri passarono dai 392 milioni di euro del 2006 ai 600 milioni del 2007, cui si aggiunsero le risorse assegnate al Ministero delle finanze e quelle destinate dal Governo all'azione di cooperazione in Afghanistan, Libano e Sud del Sudan. E con la finanziaria 2008 vi fu un ulteriore incremento, che portò a 732 milioni di euro gli stanziamenti del bilancio degli Esteri. Ciò indica con chiarezza la determinazione del precedente Governo a rispettare gli impegni assunti in sede ONU e Unione europea, impegni che prevedevano un costante aumento della percentuale di aiuto per lo sviluppo sul PIL, al fine di raggiungere l'obiettivo dello 0,70 per cento Guardando ai dati attuali sulla cooperazione allo sviluppo, bilaterale e multilaterale, è del tutto evidente che questo Governo ha compiuto solo significativi passi indietro. Infatti, i tagli al bilancio della cooperazione previsti dalla legge finanziaria 2009 hanno determinato una riduzione del 56 per cento degli stanziamenti, e l'Italia è così passata dai 732 milioni di euro del 2008 ai 312 milioni del 2009. Vedete, discutiamo spesso in quest'Aula del *corpus* giuridico delle norme che vengono approvate, del loro ancoraggio al dettato costituzionale, della loro reale efficacia ai fini del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini italiani e di chi vive e lavora in Italia; in ultima analisi, discutiamo del loro buon senso. Ebbene, in questo ambito, più di ogni altra parte, manca proprio il buon senso. Anche per questo le "perplessità e preoccupazioni" espresse dal presidente Napolitano, sulle "criticità" e la "disorganicità" nel modo di legiferare di questo Governo e della sua maggioranza, vanno - credo - accolte seriamente da tutti. Perché vedete, cari colleghi della maggioranza, avete un modo di governare che, in maniera esemplarmente lineare, risolve la necessità di nuove e tanto invocate regole della nuova economia globale e interdipendente alzando solo muri e alimentando paure e trattando da criminali proprio coloro che provengono dai Paesi ai quali avete cancellato gli aiuti. Per un Governo di un Paese del G8 che si vuole seriamente impegnare in una politica globale a favore dello sviluppo, dei diritti umani, della pace e della sicurezza c'è bisogno di strumenti finanziari adeguati. C'è bisogno di una visione complessiva e integrata della questione per essere coerenti con ciò che si sostiene non solo nei vertici europei e mondiali,

anche perché, secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il fenomeno degli "eco-profughi" è destinato a subire un aumento esponenziale: si prevede, infatti, che nel 2050 il mondo potrebbe ritrovarsi a gestire la migrazione forzata di 250 milioni di persone, con una conseguente accelerazione dei fenomeni di migrazione verso i Paesi sviluppati, e dunque anche verso l'Italia. C'è urgente bisogno di alzare il tiro, cari colleghi, non solo per consolidare credibilità d'azione nei consessi europei ed internazionali per il nostro Paese, ma perché alzare il tiro significa politiche di ampio respiro e di prospettiva futura per gli italiani, ma anche per gli immigrati, i profughi, i rifugiati, creando opportunità di pace e sviluppo nei loro Paesi e creando anche i presupposti di una solida politica dell'integrazione e della convivenza nel nostro Paese. Ecco quindi, signor Presidente, le ragioni di questa nostra mozione. Un atto politico concreto per chiedere al Governo e alla sua maggioranza di voler considerare i gravi effetti che le proprie scelte economiche hanno prodotto nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, perché, cari colleghi, oggi più che mai è necessario ricordarsi che, se Atene piange, Sparta non ride sicuramente.

non senza rappresentare il dispiacere mio personale, nonché del mio Gruppo, circa l'inopportunità di questa discussione che sarebbe stata sicuramente più utile prima dello svolgersi del G8 de L'Aquila. Oggi di fatto, colleghi, non possiamo far altro che prendere atto di ciò che il Governo ha fatto (e in troppi casi non ha fatto) in quella occasione. Proprio perché la mozione è un atto di indirizzo, sarebbe stato auspicabile discuterne in Parlamento prima che fosse posta in essere una qualsivoglia condotta da parte del Governo. Purtroppo ci limiteremo, come al solito, a discutere di ciò che è stato, con l'auspicio che in futuro, se la maggioranza dei colleghi presenti in Aula apprezzerà quanto da noi parlamentari dell'Italia dei Valori è stato riportato nel nostro documento, il Governo si ritenga impegnato a raggiungere gli obiettivi indicati. colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha volutamente escluso dal testo della mozione presentata ogni riferimento alla condotta politica e diplomatica tenuta dal Governo e, soprattutto, dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'imminenza dello svolgersi del vertice. Volutamente abbiamo evitato di inserire, tanto nelle premesse quanto nei *considerata*, passaggi circa il modo in cui il Presidente del Consiglio nel nostro Paese è solito passare la serata, in qualche lettone o con quali ragazze. Abbiamo evitato, nonostante la stampa estera e non qualche foglio comunista (ripeto, la stampa estera) avesse indicato nel *premier* Berlusconi il motivo dell'inattendibilità dell'Italia nel preparando vertice del G8 de L'Aquila. Allo stesso modo, abbiamo evitato volutamente di inserire riferimenti alle pur importanti polemiche riguardanti i costi dell'organizzazione, ai costi dello spostamento dalla iniziale sede de La Maddalena a quella finale de L'Aquila, come poc'anzi ha evidenziato Abbiamo voluto evitare di discutere di quella che comunque abbiamo ritenuto e riteniamo una spettacolarizzazione del dolore dei cittadini aquilani. Registriamo con favore che molti dei *leader* intervenuti abbiamo promesso aiuti per il recupero delle aree che hanno subito il sisma, ma voglio far presente che a L'Aquila occorreva discutere di altro e che, nonostante ciò, il fatto che si sia trattato di spettacolarizzazione è stato più volte ribadito anche in questi giorni dal primo cittadino del capoluogo abruzzese, che non mi risulta essere iscritto ad alcun partito dell'opposizione. La nostra scelta, ossia quella di voler inserire nella mozione solo elementi di discussione e di impegno riguardanti il G8, è stata una scelta sicura e consapevole, ma, visto il tenore delle mozioni presentate anche dagli altri colleghi ed il volgere degli eventi (e mi riferisco, da una parte, alla situazione disperata dei cittadini aquilani, ancora costretti in tenda e a pagare tasse ed arretrati dal 1° gennaio prossimo, e, dall'altra, al fuoriuscire di intercettazioni del *premier* Berlusconi che ci imbarazzano come italiani), ritengo più corretto parlare di quanto è stato deciso nell'appena trascorso G8 de L'Aquila e di riservarmi di esprimere eventuali considerazioni dell'Italia dei Valori sugli altri punti indirettamente connessi al G8 in dichiarazione di voto. Per ciò che attiene la mozione, dunque, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha scelto alcuni dei temi più caldi dell'agenda politica internazionale che il vertice dei Paesi più ricchi ed industrializzati avrebbe dovuto affrontare certamente con più decisione, visti i miseri risultati ottenuti. Tra questi, cari colleghi, abbiamo indicato l'ormai spaventoso problema dell'emergenza climatica e degli effetti dell'inquinamento - derivante principalmente dal consumo di combustibili fossili - sul nostro pianeta. Abbiamo inoltre scelto, per ovvie ragioni di impossibilità a citare ed esigere impegni in tutti i campi in cui si registrano purtroppo preoccupanti situazioni, di inserire nel nostro documento le difficili condizioni, soprattutto alimentari e sanitarie, in cui versano miliardi di nostri simili. Al contempo, pur essendoci limitati ad individuare queste tre macroaree di intervento, riteniamo importantissimi, anche perché troppo spesso correlati, i problemi della pace e della democrazia in alcune aree del mondo particolarmente calde in questo momento (mi riferisco all'Afghanistan ed all'Iran) ed al correlato problema della sicurezza internazionale, minacciata globalmente dal terrorismo. Venendo alla trattazione dei punti indicati nella mozione del Gruppo dell'Italia dei Valori, troviamo, nell'ordine, il grave problema del contenimento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, che contribuiscono sensibilmente al pericolosissimo riscaldamento del pianeta, il quale non permetterà il mantenimento di un equilibrio sostenibile tra le necessità di sviluppo di tutte le Nazioni e la tutela dell'ambiente. A tale riguardo, colleghi, l'Italia dei Valori denuncia una parziale sconfitta negli obiettivi che il G8 si era posto, a differenza della stragrande maggioranza dei mezzi di informazione del nostro Paese, che hanno rappresentato ai nostri connazionali, soprattutto durante i giorni del vertice, una situazione che non c'era: una falsa verità, una meschina esaltazione di risultati che non c'erano e non ci sono. Comprendiamo che, viste le premesse, le polemiche e le paure sul vertice, le televisioni e la carta stampata abbiamo potuto quanto meno tirare un sospiro di sollievo quando più di qualche importante, se non il più importante Capo di Stato straniero si è complimentato con il Governo italiano per l'ottima organizzazione del vertice. Ciò nonostante, colleghi, non possiamo che ritenere questa una magra, magrissima consolazione. I vertici del G8 - non so se è chiaro a tutti o se, peggio, non ci sia la precisa volontà di non renderlo chiaro agli italiani - si fissano, poi si organizzano e si svolgono per trovare soluzione ai principali problemi che attanagliano il nostro pianeta. Occorre svolgerli a livello di G8, forse meglio di Gl4 o, meglio ancora, di G20, perché i principali Capi di Stato e di Governo del mondo hanno il dovere di pensare non solo al benessere delle

ha inteso indicare nella mozione le gravissime condizioni in cui versano troppi esseri umani colpiti da virus e parassiti pericolosissimi quali l'HIV, la tubercolosi e la malaria. Su queste grandi emergenze sanitarie avremmo voluto che il G8 avesse proposto qualche soluzione soddisfacente, avesse quanto meno provato a chiamare per nome e cognome i problemi di cui avrebbe dovuto occuparsi, così come avremmo preferito che chi presiedeva il vertice, ovvero il nostro presidente del Consiglio Berlusconi, invece di badare ai costosi regali che imbarazzavano i suoi colleghi e a sontuose cene con o senza *first lady* al seguito, si fosse proposto almeno come ispiratore di queste improbabili soluzioni. Così purtroppo non è stato, cari colleghi, così come purtroppo non c'è stata neppure una proposta concreta e utile a sbloccare i negoziati sulle liberalizzazioni degli scambi mondiali, sconfiggendo - leggo testualmente - «il protezionismo ed adottando una carta dei principi che regoli i mercati finanziari». Si è infatti evitato di entrare in dettagli relativi alla realizzazione di detti impegni, non curandosi della grave speculazione in corso sui *futures* delle materie prime e non affrontando, anzi ignorando completamente, l'inerente problema della dannosa centralità del dollaro negli scambi mondiali. Si sono fatti solo generici accenni a non meglio specificati aiuti indicati quale soluzione del problema della fame nel mondo. Vedete, colleghi, per scrivere questa mozione, che potrà anche non piacere a qualcuno o a molti in quest'Aula, ci siamo attenuti strettamente al documento che il Governo ha pubblicato sul sito ufficiale dell'evento,

chi parla di risultati ottimi del vertice svoltosi a L'Aquila o non è informato o non ha letto i documenti o più semplicemente mente agli italiani e, considerato il tenore dei problemi in questione, mente a se stesso. Sempre nel documento ufficiale cui accennavo in precedenza è citata la ragguardevole cifra di 20 miliardi di dollari che i grandi della terra avrebbero stanziato - il condizionale è d'obbligo, cari colleghi, se si considera che la provenienza dei fondi non è nemmeno accennata - per la cooperazione allo sviluppo, ovvero per promuovere

impegna il Governo a destinare immediatamente nuovi fondi necessari al contrasto della fame nel mondo e al contrasto di malattie quali l'AIDS, la tubercolosi e la malaria; a ridurre significativamente le emissioni di gas serra (non di gas non specificati, invece nel documento approvato) nell'atmosfera; a portare soccorso ed aiuti nelle aree del mondo in cui sono ancora in corso conflitti armati; a permettere una concreta liberalizzazione dei mercati mondiali delle materie prime. Tutto ciò, colleghi, al fine di potersi presentare agli ormai prossimi appuntamenti di Copenaghen e Muskoka con una credibilità diplomatica differente, utile anche a proporre una concreta modifica del funzionamento di detti vertici internazionali, e con l'auspicio che dette modifiche che dette modifiche possano essere utili a conseguire risultati quali il miglioramento delle condizioni di vita di miliardi di esseri umani oggi in difficoltà, principalmente a causa della fame, della malattia e della guerra, oltre che della situazione climatica globale,

firmatario si concentra su uno dei tanti temi importanti che erano oggetto del vertice G8 a L'Aquila per trovare e indicare soluzioni urgenti e strutturali alla crisi economica e sociale. Il vertice G8 a L'Aquila - lo ha sottolineato il presidente D'Alia - ha rappresentato sicuramente un successo significativo per l'Italia - lo riconosciamo, lo sottolineiamo - e, ammettiamolo pure, anche per il presidente americano Obama. Il Governo italiano e segnatamente il Ministro dell'economia e delle finanze hanno promosso un processo di discussione e di confronto con gli altri Paesi membri in merito alla necessità di una riforma incisiva per il sistema finanziario ed economico internazionale in seguito alla grave crisi che continua a scuotere l'economia mondiale, provocando disoccupazione, perdita della capacità produttiva e disagio a noi tutti, ai cittadini ma, soprattutto, alle fasce più deboli anche del nostro Paese.

il Governo sui rischi inerenti ad un mercato finanziario privo di regole e di trasparenza. La prima mozione da me presentata è infatti datata 27 febbraio 2002 già in essa puntavo il dito sulle bolle finanziarie e sui rischi che comporta un liberismo sfrenato. Tutti ricordiamo le crisi finanziarie e bancarie del 1997 in Asia e in Russia, seguite poi da quella in America latina nello specifico, dal crollo della*new economy* negli Stati Uniti, oltre alla gigantesca crisi giapponese del 2002 e alla bancarotta dell'Argentina. I nostri appelli e quelli di molti altri autorevoli esperti del settore, come quello dell'economista americano Lyndon LaRouche, sono purtroppo rimasti inascoltati, con il risultato che oggi ci troviamo dinanzi ad una crisi che rischia di diventare disastrosa come quella del 1929. Oggi tutti chiedono una nuova Bretton Woods, incluso il ministro dell'economia Tremonti. Ribadisco però quanto detto prima: se qualcheduno avesse ascoltato i nostri appelli negli anni passati, avremmo potuto evitare questo disastroso crollo economico e finanziario. Ricordiamo tutti che la crisi del '29 portò la comunità internazionale a stringere gli accordi di Bretton Woods al fine di darsi delle regole precise per i mercati finanziari e valutari agli Stati fu chiesto di sorvegliare regolarmente il mercato. Ma perché, ci chiediamo, nonostante questo il sistema è andato in crisi così profondamente, e nonostante le regole di Bretton Woods? Perché all'inizio degli anni '70 si credeva di poter superare quelle regole; si credeva in un'assoluta un'assoluta possibilità dei mercati, in un liberismo totale e, soprattutto, sulla scia del liberismo americano

Ciò che è avvenuto è la mancanza di ogni forma di controllo rigoroso, l'assenza di una trasparenza dei bilanci delle società finanziarie e degli istituti di credito, nonché la mancata stabilità dei cambi valutari. Ribadisco questi aspetti perché sono importanti per capire come uscire dalla crisi. L'economia mondiale, che in passato si basava sul lavoro effettivo, sugli investimenti in infrastrutture, prodotti e servizi e, dunque, sulla creazione di ricchezza reale, si è trasformata sempre più in un'economia del debito, basata sulle speculazioni finanziarie e sulla crescita di valori fittizi. Si è fatto abuso di contratti derivati, nati, in realtà, per tutelare ed assicurare l'agricoltura, divenuti col tempo degli strumenti per realizzare, con un investimento minimo, grandi speculazioni ad altissimo rischio. Il percorso di discussione lanciato dal Governo individua una serie di principi che costituiscono la base del già citato Lecce *Framework*, adottato nella riunione dei Ministri delle finanze del G8 del 13 giugno a Lecce. Il Lecce *Framework* è stato citato nel comunicato ufficiale del G8 de L'Aquila come base per un'ulteriore elaborazione delle misure necessarie per stabilire concordemente nuove regole per l'economia mondiale, al fine di evitare il ripetersi delle pratiche finanziarie. Infatti, il processo di finanziarizzazione dell'economia mondiale, a partire dagli Stati Uniti e dai Paesi europei,

seguito da un processo di deregolamentazione che ha avuto l'effetto di spostare gli investimenti verso le attività finanziarie a breve termine e togliere sempre di più le risorse ed i capitali dalle attività più produttive. Un susseguirsi di bolle speculative, sui titoli di Stato, della cosiddetta *new economy*, e infine sui titoli ipotecari, hanno portato l'intero sistema monetario e finanziario mondiale sull'orlo del collasso. La risposta - ammettiamolo, assai tardiva - a questa crisi operata dai principali Governi si è concentrata quasi interamente sul tentativo di stabilizzare il settore bancario e finanziario - questo è il punto centrale centrale delle misure deliberate dai vari Governi - con una spesa che, tra banche centrali e iniziative legislative dei soli Paesi industrializzati, ha raggiunto la cifra sbalorditiva di decine di trilioni di dollari,

I principi enunciati nel Lecce *Framework*, indicati come provvisori e proposti come base per una discussione più ampia, si concentrano sulle regole di trasparenza per gli istituti finanziari, sull'aumento di vigilanza,

- soltanto una parte delle misure che bisognerebbe adottare per porre fine al processo di finanziarizzazione che ha caratterizzato l'economia mondiale negli ultimi decenni. Infatti, di fronte alla crisi attuale, ci sono due possibilità: attuare una correzione, inasprendo alcune delle regole per il mondo finanziario ed economico, ma senza attuare un cambiamento di fondo, di fondo, o portare quelle riforme a livello di cambiamento del sistema, rimuovendo le patologie che hanno condotto alla crisi attuale. Questo concetto è stato espresso anche dal ministro dell'economia, Giulio Tremonti, che ha chiesto un nuovo sistema «basato sull'etica». di febbraio di quest'anno (lo voglio ricordare, anche perché i *mass media* ne hanno dato poco rilievo, eppure mi pare fosse un evento importante), il Senato della Repubblica ha discusso una serie di mozioni sul tema della "nuova Bretton Woods" (si tratta, tra gli

per fermare gli effetti immediati della crisi e porre le basi per un'economia sana e non speculativa in futuro. Della nuova Bretton Woods segnalo

tasso d'interesse e a lungo termine in infrastrutture, industria e alta tecnologia. Impegniamo pertanto il Governo con questa mozione, in vista del vertice del G20 che si verrà a Pittsburgh, a portare avanti ed espandere in tutte le sedi internazionali le istanze del Lecce *Framework* per raggiungere un cambiamento fondamentale del sistema (questo il punto che vorrei sottolineare), basato sui principi della Bretton Woods. La crescita economica dovrà non più basarsi sui meccanismi speculativi come fonte di guadagno illusorio e dannoso per il benessere e la stabilità della società, ma basarsi sul progresso dell'economia reale

C'è chi dice che ci vuole un G14 e chi un G20, perché dal G8 vengono a mancare i significativi protagonisti delle economie affluenti. La stampa internazionale accorre al circo: tutti la vedono come una scena di prova per il Presidente americano, di recente elezione. Pochi si interessano alle stranezze della politica italiana e anche alle figure che farà il Presidente del Consiglio italiano. Il collega Peterlini ricordava un secondo fa che i mercati non si autogovernano, ma bisogna osservare che anche la politica internazionale non ha le idee chiarissime su che cosa si può fare e viene anche da chiedersi che, se per caso lo sapesse, questo potrebbe non essere garanzia di una efficacia effettiva. Questo il quadro di insieme in cui si muove il nostro G8 italiano, prima progettato a La Maddalena. Scanu qui ha ricordato che la cosa nasceva da una necessità di risarcimento dei danni militari in Sardegna: si spendono 320 milioni di euro per la solita urbanistica d'occasione, malattia tipica della gestione territoriale italiana (le cose si fanno soltanto quando ci sono eventi eccezionali), e poi per un motivo altrettanto eccezionale il tutto viene spostato a L'Aquila. Rispondo io alla domanda del senatore Scanu del perché è stato spostato il G8 a L'Aquila. Unicamente per una banale, enorme, colossale operazione pubblicitaria; non c'è nessun'altra motivazione.

Abbiamo assistito in onore di questa operazione pubblicitaria allo spostamento tramite ruspa delle macerie per far venir meglio le fotografie, visto la piattaforma sismica per far provare il terremoto alle signore, signore, un piccolo autoscontro assolutamente irridente verso la reale entità del fenomeno sia fisica che sociale. Vi è il problema più grave: la questione del lato

la si affronta con il solito finto decisionismo, ma non ci si chiede se la risoluzione è affidata ad analisi geologiche o ad opportunità fondiarie. Il centro storico è distrutto e si parla di *new town*, senza affrontare il problema della dispersione demografica. C'è un punto fermo: di sicuro si può continuare a fare affari. E questi affari si fanno in nome del fatto che ormai la Protezione civile, arbitra totale di tutto quel che succede in Italia negli eventi straordinari, è sottratta alla Corte dei conti. Bertolaso è plenipotenziario delegato, onnipotente ed in totale opacità ed assoluta mancanza di trasparenza. Berlusconi, con la sincerità che ogni tanto gli scappa via, dice che deve essere presente a L'Aquila perché dove dove l'occhio del padrone arriva i lavori vengono fatti meglio e la citazione, diciamo, è espressiva: l'occhio del padrone e il suo braccio. Come reagiscano i cittadini è abbastanza chiaro: si arrabbiano ed il sindaco vuole restituire la fascia tricolore. I cittadini de L'Aquila saranno costretti a pagare le tasse in modo anticipato. Insomma, stendiamo un velo pietoso su questa pena. Circa il lato politico internazionale, è un *set* televisivo, questo lo abbiamo già detto, ma va rimarcato, che il *set* televisivo è ancora una volta nelle mani della Protezione civile, che è veramente una sorta di moloch complessivo che sembra destinato a gestire tutto. Le promesse ecologiche saranno quasi sicuramente vane. Il ruolo di anfitrione del Presidente del Consiglio produce spessore politico reale solo per chi vuole vederlo a tutti costi. C'è un aspetto grottesco

cosa che farebbe sorridere se non facesse quasi piangere. Senza alcun ritegno, di fronte all'invito alla concordia proposto dal presidente Napolitano, Berlusconi ha utilizzato il suo cosiddetto successo per incrementare la polemica nei confronti dell'opposizione. Quanto varrà questo successo si vedrà. Quali e quanti fondi il Governo dedicherà alla fame lo si vedrà. Resta aperto il problema,

Resta anche un problema aperto, quello di quali e quante case e in quanto tempo saranno ricostruite a L'Aquila. Ha svettato sull'atmosfera televisiva - e non solo televisiva - da L'Aquila la questione Obama-solare-nuove energie-rifiuto dei combustibili fossili. Con coerenza ammirabile, il Governo italiano propone invece una rinuncia al solare, naturalmente realizzandola nella forma del grande elogio alla grande politica di Obama; però quando poi la grande politica di Obama pensa al solare loro al solare non pensano per niente. niente. L'unico vero successo effettivo di questo G8 è il semplice, forse un po' intorpidito, annebbiamento dello scandalo, che è errore chiamare privato: infatti, se un Capo del Governo può essere ricattato da donne a pagamento e da chi gliele procura, e perfino da soggetti terzi, che forse a proprio vantaggio possono tacere ciò che sanno, in tutto ciò non c'è l'ombra l'ombra di qualche cosa di privato. In ogni caso, comportamenti privati di questa natura invalidano nel profondo l'intera retorica del *Family* *Day* e la legge sulla prostituzione, voluta per l'appunto dall'utilizzatore finale. Il tema insomma, signor Presidente, è così triviale che rinuncio di proposito ad accenti drammatici ed abbasso i toni. Il Presidente del Consiglio, così inadatto al suo compito, si accontenti di essere l'utilizzatore finale di palazzo Grazioli; il ruolo di utilizzatore finale della Repubblica non gli si addice.

Signor Presidente, colleghi, la collega Marinaro ha prima discusso in modo approfondito i temi generali che stavano sullo sfondo del G8 condotto condotto dalla Presidenza italiana. Sono d'accordo con lei e con i colleghi che sono precedentemente intervenuti nel dire che

partecipato sarà scritta dalla storia dei prossimi anni, dal mantenimento degli impegni, dalla capacità di stare veramente nel cuore delle questioni di un mondo globalizzato; non solo dalla capacità di di interallacciare e mettere in rete tutte le nostre economie e tutte le nostre capacità di produzione e consumo, ma anche di mettere in rete le disuguaglianze, le povertà e tutta la nostra capacità tecnologica ed anche, direi, della vecchia e cara solidarietà di orientarsi nel superare queste disuguaglianze e nello sconfiggere la povertà. Nel mio intervento voglio accennare ad un punto minore del G8 che ci siamo lasciati alle spalle. Mi riferisco ad alcuni problemi organizzativi che hanno riguardato lo spostamento da La Maddalena a L'Aquila. È superata la questione dell'opportunità di tale spostamento, che noi abbiamo contestato perché non avrebbe portato a nulla, se non a qualche passeggiata ad uso delle televisioni e di una momentanea commozione dei Presidenti, dei Capi di Stato e delle *first* *lady*,cioè non avrebbe portato sicuramente niente di più in termini di volontà e di capacità organizzativa dello Stato nella ricostruzione de L'Aquila e dell'Abruzzo.

anche in questo episodio il Governo si è qualificato come un Esecutivo che non ascolta il Parlamento, che non tiene conto del suo potere di indirizzo. il 20 novembre 2008 il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adoperarsi affinché una quota delle somme stanziate per far fronte alla realizzazione delle opere del G8, allora destinate alla Sardegna, fosse quanto meno messa al riparo dalle rimodulazioni che il CIPE si apprestava a fare per la allocazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

per la ricostruzione de La Maddalena a titolo di risarcimento, ma anche a titolo di simbolo di una pagina nuova nella politica estera, per passare da un Mediterraneo

potranno essere continuate con fondi della Regione e che tutto quello che si risparmierà con i fondi della Regione potrà essere utilizzato per

per finanziare la politica estera e la politica di ricostruzione del terremoto. Sono obiettivi assolutamente legittimi e capaci di trovare merito e sostegno, ma non con questa formula che mi sembra una sorta di applicazione del principio per cui Robin Hood avrebbe dovuto, al rovescio, togliere ai poveri per dare ai ricchi. In questo caso, per soddisfare alcuni bisogni importanti si toglie ad una Regione che certamente non è ricca, caricandola di finalità generali che da sola non può sopportare.

dimostrare, ma è quello che ci aspettiamo che il Governo almeno tenti di fare, in risposta alla mozione. Sempre con la mozione, chiediamo che si utilizzino le strutture realizzate in Sardegna per vertici internazionali, che possano in qualche modo "risarcire" la

Sarebbe un vero e proprio sviamento nell'opera di allocazione delle risorse che democraticamente la Regione ha deciso di operare sulla base di presupposti del

Signor Presidente, la legge n. 146 del 1990 prevede che i membri della Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici siano nominati dal Presidente della Repubblica, su designazione congiunta dei Presidenti delle Camere. Poiché l'atto di nomina del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Ministro del lavoro, è quest'ultimo a risponderne sul piano politico, a norma dell'articolo 89 della Costituzione, ed è proprio questo il motivo per cui, il 7 luglio scorso, ho presentato alla Presidenza del Senato un'interrogazione su questa materia, rivolta appunto al Ministro del lavoro, segnalando le incongruenze delle designazioni che risultano essere state proposte ultimamente dai Presidenti di Camera e Senato, rispetto ai requisiti posti dalla legge citata, per i membri della Commissione di garanzia, e chiedendo come il Ministro stesso intendesse procedere per risolvere questa questione. del Senato mi ha comunicato, con lettera protocollo n. 3372/S, di non ritenere ammissibile quella interrogazione per difetto di competenza del Governo. Ora, poiché evidentemente non è pensabile che su una questione tanto delicata sia precluso al Senato di discutere, non mi resta che chiedere a lei di riferire in quest'Aula circa i criteri seguiti nella designazione in questione e di consentire che in questa stessa sede la questione venga discussa apertamente. Mi rendo conto della difficoltà costituita dall'assenza di precedenti parlamentari in materia, ma la delicatezza e l'importanza della questione impongono che da questa *impasse* determinatasi si esca con scelte che siano il risultato di un dibattito aperto e del tutto trasparente. La ringrazio dell'attenzione e resto in atteso delle sue determinazioni.

che di questo argomento non se ne doveva neppure parlare, anche perché si fa riferimento a valutazioni che riguardano proposte e decisioni dei Presidenti delle Camere e del Presidente della Repubblica.

ha comunque detto, con riferimento alla sua interrogazione, che era inammissibile. Questo è lo stato dell'arte; in ogni caso, prendo atto delle sue dichiarazioni. accetto la dichiarazione di inammissibilità dell'interrogazione, anche se non ne condivido la motivazione, perché la Costituzione afferma

ci sarà pure il modo di discutere di questo atto politico

che si possono anche cambiare, per carità; magari suggerisca lei il modo, dal punto di vista parlamentare, per poterlo fare. **Sull'assenza

leggere alcuni commi del nostro Regolamento, che tutti noi rispettiamo, meno, da un anno a questa parte, il Consiglio di Presidenza, il Presidente del Senato e tutti i suoi componenti.

«Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione

«il Presidente ne riforma il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati». Ora mi chiedo, e si chiede il mio Gruppo (lo ripeterò ogni giorno

che cosa ha riferito il Presidente del Senato sul fatto che è stato composto un Consiglio di Presidenza monco del quarto partito in Italia, secondo partito del centrosinistra,

«sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato». E l'Italia dei Valori è da un anno assente in questa sede. L'articolo 11 del Regolamento recita: «I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete»

«vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza...». Ma quel che fa maggiormente indignare, per quanto riguarda il nostro Gruppo dell'Italia dei Valori, signor Presidente, «Il Consiglio di Presidenza (...) delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo;». E noi non ci siamo: non abbiamo votato, perché non c'eravamo, e non abbiamo potuto interpretare cosa è stato detto durante il dibattito, perché

articolo 12, «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;». Il personale si sta lamentando di avere

dando le deleghe piene come le avete date agli otto Segretari d'Aula presenti da un anno. Noi non siamo presenti ed oggi siamo orgogliosamente qui a protestare per la legittimazione di una presenza che il Regolamento del Senato richiede. Ma se la richiede il Regolamento del Senato, mi spieghi il Presidente del Senato perché da un anno avete cancellato

Per quanto riguarda la sua espressione riferita al Segretario generale, lei sa che il Segretario generale è il Segretario generale del Senato e non del Presidente. Peraltro, le ricordo che l'attuale Segretario da questo Presidente del Senato.